riguardante la manifestazione dei liberi professionisti, probabilmente andrebbe aggiunto che essi non si sono limitati ad intervenire, ma hanno chiesto una risposta da parte del Governo e c'era stato anche il suo impegno personale a far sì che il Governo rispondesse. Credo che di questo debba essere lasciata traccia nel processo verbale.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità alcune limitate modifiche ed integrazioni al calendario corrente, già comunicato all'Assemblea, con l'intesa che la Conferenza sarà riconvocata martedì 24 ottobre alle ore 9 per la definizione del calendario a partire dal 7 novembre. Questa mattina, dalle ore 10,30 - per consentire ai senatori della 4a Commissione permanente di assolvere ad un impegno internazionale - inizierà la trattazione del decreto-legge sulla missione in Libano, che dovrebbe concludersi in giornata. quindi bisogno di una breve sospensione la faremo fino alle 10,30. Resta poi confermato per questa settimana, con eventuale seguito nella prossima, l'esame dei decreti-legge in materia di intercettazioni telefoniche (quest'ultimo con inizio domani mattina) e in materia di disagio abitativo, nonché dei disegni di legge recanti rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato e degli altri argomenti già previsti dal calendario. Nella seduta antimeridiana di giovedì 19 ottobre saranno rese all'Assemblea le comunicazioni del Presidente sul disegno di legge collegato in materia di servizi pubblici locali. Nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre il *question time* sui diritti umani in Cina avrà luogo con trasmissione diretta televisiva. Si aggiunge inoltre per la settimana prossima la discussione della mozione Mantovano ed altri sui flussi migratori. colleghi, occorre procedere all'avvicendamento tra un componente effettivo e un componente supplente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa-UEO.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Sulla base delle designazioni del Gruppo interessato, il Gruppo Misto, il senatore Barbato e il senatore Formisano - entrambi già facenti parte della delegazione

un episodio molto grave, ci sono tantissime ambulanze che si stanno recando presso la stazione Vittorio Emanuele della metropolitana di Roma; credo sia importante che il Parlamento venga messo a conoscenza di quanto è accaduto.

Presidente, ci associamo pienamente alla richiesta del senatore Storace. Anche noi senatori del centro-sinistra siamo in paziente, ma trepidante attesa di avere informazioni su questo grave incidente che non ha precedenti precedenti nella città di Roma. Siccome molti di noi, come il senatore Storace, hanno a cuore non solo i cittadini ma la realtà della città, la preghiamo cortesemente di sollecitare, con grande vigore e forza, il Governo affinché ci fornisca le informazioni che ha chiesto il senatore Storace.

Vorrei però intervenire su un'altra questione che credo non sia secondaria, e cioè su quanto sta accadendo in questo momento in Senato relativamente alla libertà di esercizio delle funzioni dei singoli senatori. È noto a tutti che la Giunta delle elezioni sta esaminando un caso assai delicato, ossia il ricorso dei candidati del partito della Rosa nel Pugno,

evidente e normale, se ne sta occupando la Giunta delle elezioni e ne è stato nominato relatore il senatore Manzione, il quale, venerdì 13 ottobre, ha emesso un comunicato stampa che credo debba essere considerato attentamente, non soltanto dalla Presidenza, ma, stante la gravità della questione, da tutta l'Assemblea che quindi ne deve essere edotta. ne deve essere edotta. Da quanto si evince dal comunicato emesso dal senatore Manzione, sembrerebbe che il senatore stesso avesse avuto l'intenzione di esprimere pubblicamente la sua convinzione - che evidentemente nasce dall'esame degli atti e degli esiti delle votazioni, non certo da considerazioni politiche - secondo la quale alcuni ricorsi non erano manifestamente infondati. lui stesso dichiara che il suo comunicato è stato bloccato e che il senatore Zanda, brandendo la nota, con tono minaccioso, si è scagliato contro di lui.

esercitare le sue funzioni ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, e questo fatto è ancor più grave perché il senatore Zanda è parte in causa in quanto perderebbe il seggio nel caso in cui il senatore Manzione o la Giunta decidessero in un certo modo. Credo sia un fatto di una gravità inaudita e la prego, Presidente, di prenderlo in esame.

si introducono argomenti risibili che non rispondono assolutamente al vero e si apre una questione, anche un po' disdicevole, che non trova assolutamente riscontro nella realtà dei fatti, tra l'altro, con un'ingerenza nella vita degli altri Gruppi che non riguarda assolutamente il Gruppo della Lega e il collega Castelli. Presidente, qui non possiamo ogni volta

Senatore Boccia, non si apre alcuna questione. Se ci sono questioni da approfondire lo faremo, ma ho già risposto al senatore Castelli che doveva stringere perché non si può aprire nessuna discussione su questo punto; c'è la Giunta delle elezioni che sta lavorando. Per quanto riguarda l'incidente alla metropolitana di Roma, mi associo alle preoccupazioni dei senatori intervenuti. Ci attiveremo immediatamente affinché il Governo venga a fornire le delucidazioni richieste dal Senato.

e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, cominciamo oggi l'esame del disegno di legge n. 1026, già approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, che converte in legge, con modificazioni, il decreto n. 253 con cui il Governo ha disposto, il 28 agosto scorso, l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 2006 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E' stata già oggetto di un ampio dibattito politico la decisione di un impegno di primo piano del nostro Paese, nello sforzo della comunità internazionale, teso in primo luogo a mettere fine alle ostilità che hanno fatto tante vittime e arrecato così gravi danni alle infrastrutture civili in Libano e in alcune città della parte settentrionale di Israele; e teso a rimuovere, con la collaborazione dei due Stati sovrani coinvolti nella guerra, Israele e Libano, le cause ormai antiche e strutturali che hanno portato al riesplodere del conflitto. Il dibattito politico ha rilevato un orientamento pressoché unanime del Parlamento a sostegno della missione, sia con la risoluzione del 18 agosto delle Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato, sia con il voto della Camera che ha approvato il disegno di legge il 26 settembre. Mi preme qui sottolineare come la responsabile, ampia e consapevole convergenza del Parlamento, sollecitata fin da agosto dal Governo, abbia avuto un ruolo decisivo sia nell'aiutare il nostro Governo nella complessa trattativa internazionale che si è svolta per decidere della composizione della missione e delle sue regole di ingaggio, sia nel creare un clima di condivisione della stessa nell'opinione pubblica del nostro Paese. Voglio ricordare che il primo voto del Parlamento, espresso il 18 agosto, ha rafforzato l'autorevolezza e la credibilità della posizione italiana in giorni in cui non era ancora affatto chiaro se altri importanti paesi europei, la Francia in primo luogo, sarebbero stati disposti a un impegno analogo. Si è trattato di una buona prova di serietà sulla scena internazionale e di consapevolezza dell'interesse nazionale, che mai come in casi di missioni militari all'estero merita di essere preposto alle differenze e alle polemiche politiche tra maggioranza e opposizione. La risoluzione 1701 dell'ONU, e la disponibilità subito dichiarata dal nostro Paese di darle seguito rafforzando con proprie truppe la missione UNIFIL, ha avuto un primo rilevante effetto: ha ottenuto un cessate il fuoco che dura tuttora e ha dunque fermato il conflitto e con esso la carneficina. Ora la missione UNIFIL è chiamata a collaborare con il Governo del Libano, sul cui territorio opera, per dare attuazione a quei punti della risoluzione 1701 che intendono rimuovere le cause del conflitto. Il più rilevante tra questi è sicuramente la restaurazione della piena sovranità del Governo di Beirut sul sud del Paese; ciò fornirebbe, di conseguenza, garanzie di sicurezza ad Israele, che da quella parte del territorio libanese aveva subito l'attacco delle milizie Hezbollah cui ha risposto con la guerra e l'invasione. In questo senso la missione UNIFIL funge davvero come forza di interposizione, neutrale rispetto alle parti in conflitto ma non neutrale rispetto alle cause che hanno provocato il conflitto. Su questo punto, che è il più controverso e anche quello che più ci preoccupa, credo che la risoluzione 1701 sia più chiara di quanto si dica, almeno nelle sue finalità. Essa prescrive infatti all'articolo 8 l'istituzione, nella zona compresa tra la Linea Blu e il fiume Litani, di un'area priva di personale armato, di posizioni e di armi che non siano quelle dell'esercito libanese e delle forze UNIFIL; la piena attuazione di tutti i Regolamenti previsti dagli accordi di Taif e dalle risoluzioni 1559 del 2004 e 1680 del 2006, che impongono il disarmo di tutti i gruppi armati in Libano, in maniera tale che non possano esserci armi o autorità in Libano se non quelle dello Stato libanese; l'istituzione di un embargo internazionale sulla vendita di armi e materiali dal Libano. La risoluzione aggiunge al paragrafo 11 che la missione UNIFIL «... assiste le forze amate libanesi in operazioni mirate alla definizione dell'area prevista nel paragrafo 8». Sul come questo processo di progressivo smantellamento delle milizie armate libanesi possa avvenire mi rifarò alle parole che il ministro D'Alema ha usato nel dibattito alle Commissioni riunite esteri e difesa della Camera, il 6 settembre scorso: «L'impianto della risoluzione delle Nazioni Unite è che il disarmo di Hezbollah sia il risultato dell'azione politica e militare del Governo libanese stesso, assistito dalla comunità internazionale e dall'UNIFIL. Questo evidentemente significa che la forza UNIFIL non ha il mandato di disarmare direttamente Hezbollah, ma ha il mandato di contribuire e rendere possibile questo risultato». Nella riunione delle Commissioni esteri e difesa del Senato, il ministro della difesa Parisi ha poi precisato che, pur essendo coperti dal necessario riserbo i dettagli delle regole di ingaggio riguardanti i militari i militari italiani, questi hanno in Libano la possibilità di esercitare l'autodifesa proteggendosi adeguatamente o utilizzando la forza in modo proporzionale alle circostanze in caso di attacco o anche nel caso di imminente attacco. Le regole adottate prevedono che sia consentito l'uso della forza contro chiunque tenti di impedire ad UNIFIL di espletare i propri compiti o tenti di limitarne la libertà di spostamento. È consentito l'intervento attivo anche nel caso sia messa in pericolo l'incolumità della popolazione civile e, concludeva il ministro Parisi, la dinamica di un eventuale incontro nella propria area di competenza di unità UNIFIL con personale armato non facente parte delle forze regolari libanesi passerà quindi - qualora le circostanze lo consentano - attraverso le fasi di identificazione, di intimazione a deporre le armi e a sottoporsi agli accertamenti necessari, di sequestro di tutti gli armamenti indebitamente detenuti e di eventuale detenzione del personale coinvolto; in tutte queste fasi sarà determinante il ruolo svolto dagli ufficiali di collegamento libanesi. Come vedete, si tratta di un compito difficile e in una zona di operazioni ad alto rischio, ma vale la pena provarci. Si è aperta una finestra di opportunità in Libano, causata anche dall'estenuazione dei due contendenti. Israele che, per la prima volta nella sua storia, ha accettato di affidarsi alla protezione della comunità internazionale dopo una guerra intensa che non ha raggiunto i risultati strategici che si proponeva, e cioè il disarmo forzato di Hezbollah. E il Libano, speriamo consapevole che la sua giovane democrazia non ha un futuro di pace e di prosperità se non si riappropria di una piena sovranità statuale e se lascia che a decidere del suo destino, della pace e della guerra, siano le milizie armate di questo o di quel partito. Auspichiamo, dunque, che il Governo Siniora ripaghi il sostegno della comunità internazionale, con la disponibilità ad avviare colloqui di pace con il Governo di Israele. La risoluzione 1701, comunque la si legga, si basa infatti su due ritiri: il ritiro dell'esercito di Israele al di là della Linea Blu, ormai completato, e il ritiro della milizia in armi di Hezbollah dal sud del Libano, sulla cui frontiera è ormai arrivato, dopo quarant' anni di assenza, l'esercito regolare libanese. La missione UNIFIL 2 continua dunque a prospettarsi come «lunga, impegnativa, costosa e rischiosa», secondo l'espressione del ministro Parisi, ma allo stesso modo appare necessaria. Essa corrisponde all'interesse nazionale, perché l'Italia e tutta l'Europa mediterranea hanno un interesse diretto e particolare alla stabilità dell'area mediorientale. E si avvale di un clima generale nei rapporti interni alla comunità internazionale anch'esso nuovo e proficuo. Lo sforzo comune sul Libano sta infatti mostrando i tratti di un «multilateralismo efficace», un multilateralismo con i denti, che non si limita cioè a chiacchierare ma agisce; che non esclude l'uso della forza militare ma la mette al servizio di una politica e di un'azione diplomatica e umanitaria. Grazie a una nuova intesa tra Stati Uniti ed Europa, in cui il Governo italiano ha sicuramente svolto un ruolo da protagonista, tutti i fori multilaterali sono impegnati in Libano: il Consiglio di sicurezza dell'ONU e l'Unione Europea in primo luogo. Decisiva sarà la fermezza nei confronti dei paesi che hanno finora svolto un ruolo negativo nel conflitto, come la Siria e l'Iran, cui viene offerto di partecipare da attori responsabili nell'attuazione della risoluzione 1701, ma a cui viene chiesto di non ostacolare la missione UNIFIL, soprattutto collaborando a fermare i commerci di armi, cosicché non ci sia un riarmo di Hezbollah lì dove dovrebbe esserci disarmo; e decisiva sarà la ripresa di un dialogo israelo-palestinese per la soluzione di lungo termine della madre di tutti i conflitti mediorientali. In entrambi i sensi il Governo italiano si sta adoperando con impegno nei confronti del mondo arabo, anche utilizzando il credito che presso quel mondo ha assunto e che - nel suo nuovo ruolo di membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU -può risultare prezioso, ai fini della costruzione di un'entità statuale per i palestinesi e della integrità e sicurezza di Israele, entrambi punti cardine della politica estera dell'Italia e dell'Europa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le Commissioni esteri e difesa hanno dato ai relatori il mandato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. Nel dibattito si è registrata un'ampia convergenza sulla necessità che il nostro Paese svolga una politica estera attiva, nel quadro delle iniziative delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, per la costruzione di un ordine internazionale di pace e la consapevolezza che l'utilizzo in missioni internazionali delle nostre Forze armate è l'adeguata proiezione di una tale politica estera, soprattutto laddove un progressivo decadimento della sovranità di alcuni Stati arreca instabilità, più che mai quando questo accade in aree geografiche che rivestono un'importanza cruciale per la sicurezza e la pace nel Mediterraneo. Le Commissioni hanno anche manifestato un ampio consenso nell'esprimere sostegno e solidarietà alle nostre Forze armate, impegnate in tutte le missioni internazionali di pace in corso, nel rispetto dei valori dell'articolo 11 della Costituzione. Auspico, quindi, che il Senato possa approvare a larga maggioranza il provvedimento, così come è avvenuto alla Camera dei deputati.

Presidente, onorevoli senatori, sostituisco nel ruolo di relatore il senatore Ramponi, cui rivolgo i miei auguri per una spinosa questione familiare che gli impedisce stamane di rappresentare in quest'Aula la Commissione difesa nella discussione del disegno di legge sull'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e di rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL. Un clima di condivisione e di solidarietà alle nostre Forze Armate impegnate nella delicatissima missione di pace in Libano ha permeato l'esame del provvedimento nella sede istituzionale delle Commissioni riunite esteri e difesa. La sintesi di quest'atmosfera di responsabilità politica ed istituzionale sarà, mi auguro, il *leit motiv* della discussione di quest'Aula, che si appresta, attraverso la conversione in legge del decreto-legge, a segnalare che sui grandi temi della politica estera e sui nostri militari, portabandiera nel mondo di un'identità solidale che costruisce la pace e contrasta la rete di morte del terrorismo integralista, la politica ritrova larghe intese e soluzioni *bipartisan* che rafforzano l'immagine internazionale del Paese. Non è un caso che proprio il senatore Ramponi abbia aperto la sua relazione in Commissione difesa, riconoscendo al ministro degli affari esteri Massimo D'Alema di aver sviluppato un grande lavoro d'interposizione fra le parti in causa nel conflitto Israele-Hezbollah, rendendo l'Italia protagonista di una mediazione di pace fra le parti, che eleva il nostro prestigio nel ruolo della costruzione della pace e porta il risultato di una maggior sicurezza al contingente impegnato in questa delicatissima missione. Va riconosciuto un dato forte, sul quale la condivisione delle scelte diventa cemento per questo ulteriore atto di responsabilità delle forze parlamentari: che missione di pace è questa del Libano e missioni di pace erano quelle nelle quali il Paese era stato impegnato negli anni scorsi su richiesta e mandato delle Nazioni Unite. Non c'è discontinuità politica che tenga dinanzi a questa onesta e necessaria considerazione. Personalmente, credo e sono certo che proprio in questo caso, evocato come rischioso e difficile, la pace, invece, durerà in forza di alcune considerazioni che sono state analizzate nel corso del dibattito in Commissione difesa. La certezza mi viene dal fatto che Israele, provocato in una reazione militare dal sequestro di due suoi militari, ha preso atto, dopo settimane di bombardamenti, che la forza di Hezbollah non è soltanto un problema regionale. Hezbollah, partito politico e forza militare, vive del sostegno concreto di Paesi terzi, l'Iran in particolare, che sarebbe un errore escludere dal tentativo di costruire la pace in quell'area. Se una manifesta assenza indebolì il vertice di Roma sul Libano quando ancora infuriava il conflitto, fu proprio quella di Iran e Siria che al Governo italiano hanno espresso la volontà di accettare una mediazione europea permanente, affidata proprio al nostro Paese, primo *partner* commerciale in particolare dell'Iran, con cui bisogna accettare di dialogare nel segno della diplomazia e della sicurezza internazionale. La missione in Libano certifica da parte nostra ad Israele l'impegno dell'Italia nella tutela della sicurezza di quel Paese. L'intervento del collega Ramponi certificò al ministro D'Alema, nonostante le molte critiche, il dato dell'intuizione di un percorso positivo che non poteva e non dovrà escludere alcuna delle parti interessate dal confronto che dovrà rendere stabile e duratura la tregua. Se Israele ha accettato la mediazione internazionale e dell'Italia in particolare sullo scambio dei prigionieri, trattativa che porterà a casa i due militari israeliani rapiti da Hezbollah, in cambio di ben nove capi politici libanesi, sul cui rilascio l'Iran farà da parte mediatrice, allora vuol dire che le condizioni per allontanare il rischio di una ripresa del conflitto si stanno costruendo e che la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha restituito voce alla diplomazia e ad al confronto. Durante il dibattito in Commissione difesa si è discusso a lungo di uno dei problemi principali della missione, il disarmo di Hezbollah. Hezbollahdovrà integrarsi nella vicenda politica e militare libanese e si tratterà sicuramente di un percorso difficile e complesso. La comunità internazionale e la stessa risoluzione delle Nazioni Unite si pronunciano nel senso della responsabilità di quel Governo e di quell'esercito che - è vero - è permeato da 13.000 soldati sciiti e da ufficiali simpatizzanti di Hezbollah, con il quale il contingente UNIFIL dovrà collaborare, ma che dovrà prendersi carico di questo percorso, un percorso che tuttavia prevarrà sulla logica della contrapposizione armata, poiché anche questa volta sarà la diplomazia a farla da padrone e a trionfare. II pericolo per il nostro contingente, anche in Libano, proverrà come altrove dalla rete di morte di Al Qaeda che ha stretto un patto transnazionale con piccoli movimenti integralisti che dal Medio Oriente all'Afghanistan, dall'Islam africano all'Estremo Oriente, hanno costituito un sistema che punterà a dimostrare che destabilizzando gli equilibri della pace si allontana l'Occidente dai Paesi che l'integralismo intende permeare. L'irachizzazione del conflitto afgano, l'utilizzo dei kamikaze, singolare per quell'area, contro i contingenti militari delle Nazioni Unite, interesserà probabilmente anche il Libano, dove alcune fazioni minoritarie puntano a creare il caos e a destabilizzare lo stesso Governo libanese. Lo dicono le valutazioni di rischio dei servizi di sicurezza europei, che in queste aree stanno svolgendo uno straordinario compito di prevenzione ed è da questa minaccia principale che dovremo difenderci. Sostenere che andando via, aprendo il dibattito sull'opportunità di riportare a casa i nostri contingenti, si risolva ogni problema di rischio è quasi un'oscenità politica. Anzi, al contrario, se il terrorismo integralista comprenderà che attaccando i nostri militari si velocizzeranno i tempi di uscita dai Paesi in cui siamo impegnati, allora sì che il tiro al bersaglio sul contingente italiano diventerà la regola.

un'ultima considerazione. Votiamo per il rifinanziamento della missione in Libano partendo da concezioni politiche sicuramente diverse, sulle quali in tema di difesa spesso è difficile perfino intendersi. Su un solo valore credo che questa volta prevalga il senso comune della responsabilità: la solidarietà verso le Forze Armate, che devono sentire il Paese vicino e forte nella volontà di rafforzare il ruolo umanitario dell'Italia,

La seduta è ripresa.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il Ministro della difesa avrebbe avuto forse il dovere di essere oggi presente insieme al Ministro degli esteri, visto che

Il Ministro della difesa ha definito questa missione lunga e rischiosa. Il Presidente del Consiglio ha vantato il ruolo di avanguardia, sostenuto dall'Italia, nella decisione di inviarla e se ne è dunque assunta la responsabilità.

di continuo. MALAN *(FI)*. La comunità internazionale e le parti in causa ci hanno richiesto questo impegno ed hanno espresso gratitudine perché l'abbiamo preso. Noi dell'opposizione, proprio perché ne conosciamo le difficoltà, abbiamo in gran parte deciso di appoggiare la missione in risposta alla comunità internazionale per evitare che, per quanto sta a noi, la missione diventi di parte e, dunque, ancora più rischiosa. Andrebbe ricordato che la stessa cosa si poteva dire della missione in Iraq. Era una missione rischiosa, fatta su richiesta e su mandato delle Nazioni Unite, il cui Segretario generale ha più volte ringraziato l'Italia per avervi preso parte e con il consenso delle parti in causa: la coalizione che ha condotto la guerra, da una parte, e il Governo iracheno, dall'altra, prima quello provvisorio e poi quello democraticamente eletto dal popolo iracheno. Ci è solo mancato il consenso del deposto Governo criminale di Saddam Hussein e dei terroristi che, oltre fare vittime tra i soldati della coalizione, fanno strage di pacifici cittadini iracheni; così come oggi la missione dell'ONU in Libano non ha il consenso dei terroristi di Al Qaeda che hanno già diffuso le loro minacce. Ebbene, sull'Iraq il centro-sinistra non ha mai smesso, neppure oggi che è al Governo, di strumentalizzare, di polemizzare e di accusare il Governo Berlusconi, arrivando all'esplicito falso, affermando cioè che l'Italia in Mesopotamia ha partecipato alla guerra. Questa falsa affermazione l'ha fatta persino in quest'Aula, per bocca del Presidente del Consiglio, - a quanto pare - il senso di responsabilità è come il coraggio: chi non ce l'ha non può darselo. Il fatto che noi invece ce l'abbiamo è una delle ragioni del consenso che ci danno i cittadini non irregimentati e meno influenzabili dalle parole d'ordine e dagli *slogan* di piazza. Che le missioni in Iraq e in Afghanistan siano missioni di pace è certificato anche dall'assenso dei Presidenti della Repubblica, prima Ciampi e poi Napolitano, che mai avrebbero potuto autorizzare una violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Pertanto, a mio parere, poiché la realtà dei fatti è evidente, quel discorso è chiuso. Ora è importante parlare del futuro perché migliaia di nostri militari sono oggi in Libano; è responsabilità innanzi tutto del Governo e della maggioranza dare alla missione un assetto politico e operativo che ne attenui, per quanto possibile, i rischi e che impedisca che questi rischi siano inutili. È responsabilità del Parlamento, in particolare dell'opposizione, che non ha espresso - né in generale ha - fiducia in questo Governo. È dunque compito dell'opposizione dare il suo contributo anch'essa in tal senso. La missione UNIFIL ha origine dalle risoluzione delle Nazioni Unite del 19 marzo 1978 che aveva lo scopo, nel breve termine, di confermare il ritiro delle truppe israeliane e, nel lungo termine, cito la risoluzione, di assistere il Governo del Libano nell'assicurare il ritorno alla sua effettiva autorità nel Sud del Paese, dove già allora imperversavano le milizie armate non governative. Il primo obiettivo fu rapidamente raggiunto, il secondo attende ancora oggi la sua realizzazione, benché richiesto, ricercato e invocato in numerose altre risoluzioni, e nonostante la decennale presenza della missione internazionale che ha anche subito pesanti perdite. Il fallimento nello stabilire un'autorità statale in Libano, soprattutto nel Sud, dovuto ad una complessità di cause, ha determinato a sua volta una permanente instabilità della zona e lo scoppio, a più riprese, di aperte ed ampie ostilità. Con il passare degli anni, il ruolo delle milizie è anzi diventato sempre più importante, tanto che le Nazioni Unite sono passate a citarle espressamente; la risoluzione 1559 del settembre 2004 chiese, infatti, lo scioglimento e il disarmo delle milizie libanesi e non libanesi. Nella risoluzione 1655 del 31 gennaio di quest'anno si menziona specificamente Hezbollah come iniziatore delle ostilità e autore del lancio di missili su Israele. Ancora la risoluzione 1680 del 17 maggio scorso nota che lo scioglimento delle milizie non è ancora avvenuto, pur apprezzando che il dialogo nazionale libanese abbia deciso il disarmo delle milizie palestinesi fuori dai campi dei rifugiati entro sei mesi. Non è un caso che in questa situazione le ostilità siano riprese. La stessa risoluzione 1701 ricorda che ciò è avvenuto a seguito dell'attacco di Hezbollah a Israele il 12 luglio. Tutto questo ci ricorda che, se non ci sono progressi sui punti principali della risoluzione 1701 e delle risoluzioni precedenti, neanche la missione ampliata, oramai in corso, potrà avere successo e dunque rischierà di ritrovarsi in mezzo a nuove ed aperte ostilità. Da quando, in agosto, il Governo si è impegnato nella questione libanese, abbiamo avuto, pur nel nostro atteggiamento di collaborazione, più di un motivo di preoccupazione. Ci ha preoccupato la passeggiata del Ministro degli esteri sottobraccio a esponenti di Hezbollah che pochi mesi prima, da parlamentare europeo, aveva, in un voto ufficiale, incluso tra le organizzazioni terroristiche *(Applausi dal Gruppo FI)*. Ci hanno preoccupato le reiterate e pesanti critiche da parte dello stesso ministro D'Alema - purtroppo oggi assente - nei confronti di Israele e degli Stati Uniti, alle quali, nonostante la proclamata equivicinanza, non hanno fatto riscontro critiche, almeno analoghe, nei confronti della controparte. In particolare, l'onorevole D'Alema ha più volte dichiarato che la reazione di Israele sarebbe stata sproporzionata agli attacchi ricevuti. Ebbene, si dà il caso che proprio il capo di Hezbollah, il signor Hassan Nasrallah, abbia affermato il contrario. Infatti, in un discorso ai suoi militanti, riportato integralmente e senza commenti dal sito Internet dell'UCOII (e di questa organizzazione contigua a organizzazioni terroristiche occorrerà parlare in quest'Aula), in quest'Aula), Nasrallah si vanta di aver inferto al nemico - cioè Israele - danni assai più pesanti di quelli subiti. Pertanto, ministro D'Alema assente, la proporzione c'era e come, per ammissione dello stesso avversario d'Israele. Ci ha preoccupato la visita del presidente Prodi in Medio Oriente, perché, dopo aver incontrato - com'è giusto - le nostre truppe, ha pensato bene di incontrare le autorità libanesi, ma non quelle israeliane; ed agli stessi soldati israeliani ha ricordato l'importanza della loro missione per l'ONU, per l'Unione Europea e per il Libano, dimenticando Israele, sul quale, dall'area dove oggi si trovano i soldati, due mesi fa piovevano migliaia di missili, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le loro case. *(Applausi dal Gruppo FI).* Oggi questo non succede più, grazie anche ai nostri soldati. Ci preoccupano le dichiarazioni del capo di Hezbollah nel Sud del Libano, Nabil Kauk, il quale afferma tranquillamente, secondo quanto si legge sul «Corriere della Sera», che Hezbollah mantiene e manterrà le armi anche a Sud del fiume Litani e che continua a riceverne dal confine siriano, come risulta anche da varie fonti giornalistiche. Più di tutto ci preoccupa l'atteggiamento generale del Governo, che sembra a volte preoccupato più di compiacere Hezbollah che di adempiere al mandato delle Nazioni Unite. *(Applausi dal Gruppo FI).* E questo non solo perché non abbiamo simpatie per un'organizzazione come Hezbollah, strumento della parte più estremista del regime iraniano, che usa la religione come giustificazione e fine della violenza armata, il cui capo arringa la folla esortando a ripetere uno *slogan* declamato da anni, «morte all'America». La questione più importante, però, è che un atteggiamento del genere non consentirà di compiere progressi verso una pace duratura, come invece ci chiedono di fare le Nazioni Unite. Un atteggiamento di compiacenza nei confronti di una delle due parti, quella apertamente violenta ed aggressiva, può dare, sì, l'illusione di allontanare il pericolo, ma in realtà incoraggerà questo soggetto a farsi più aggressivo e dunque a creare, in ogni caso, un pericolo per l'area. Per questo motivo, diversi colleghi ed io abbiamo presentato un ordine delgiorno

di esaminare con equanimità. In tale ordine del giorno non abbiamo fatto altro che riportare i punti principali della risoluzione 1701, così come sintetizzati nel paragrafo 8 della stessa, chiedendo al Governo italiano di operare con tutti i mezzi a sua disposizione - perché naturalmente non dipende solo dall'Esecutivo - per la loro piena implementazione e di riferire regolarmente al Parlamento sul livello di raggiungimento degli obiettivi, in particolare di quelli mai raggiunti prima.

nel medio termine inutile e sempre più pericolosa: dunque, dovremo comportarci di conseguenza. Confidiamo che il Governo voglia accogliere l'ordine del giorno in esame in quanto la nostra leale collaborazione, anche critica, quanto serve. I nostri soldati per primi sanno che saremo sempre vicini e solidali con loro in ogni circostanza.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole al provvedimento in esame ed auspico che, come già avvenuto nelle Commissioni riunite esteri e difesa, anche in quest'Aula si realizzi il più ampio consenso sulla missione italiana in Libano. Le motivazioni di fondo che spiegano il ruolo particolarmente attivo svolto dal nostro Paese fin dai primi segnali della crisi sono da ricondurre all'importanza geostrategica del Medio Oriente e della sua stabilità per la sicurezza dell'Europa e dell'Italia; all'esigenza di contribuire, definire ed attuare quel multilateralismo efficace di cui è esempio concreto la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, che deve orientare l'approccio della comunità internazionale nella gestione e soluzione delle crisi; e, in ultimo, alla volontà di sostenere un nuovo ruolo politico e strategico dell'Europa nella Regione medio-orientale. Nell'argomentare le motivazioni che sostengono la scelta di un voto favorevole al disegno di legge di conversione, però, credo si possano effettuare alcune osservazioni, partendo da un'analisi lessicale dell'oggetto stesso del provvedimento e che ritengo rivestano anche, e soprattutto, carattere sostanziale. Le disposizioni, si legge nel titolo, concernono l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano ed il rafforzamento del contingente militare italiano. È un'importante inversione culturale e politica, l'idea che il processo di pace possa ottenere dei risultati non soltanto dal consolidamento della tregua e dall'avvio di un negoziato politico, ma anche dalla ricostruzione del Libano e da un'azione umanitaria che la comunità internazionale deve condurre a sostegno della popolazione civile ed insieme al Governo libanese. È questo un modo efficace per non lasciare spazio solo all'azione umanitaria di segno islamista, già ampiamente avviata, che potrebbe aggravare i rischi di un ampliamento del consenso alle posizioni politiche più integraliste, poiché l'assistenzialismo è una delle forme più diffuse di proselitismo radicale. Credo siano quindi anche ragioni politiche e non solo di carattere umanitario, sicuramente non secondarie, a richiedere un intervento della comunità internazionale e, segnatamente del nostro Paese, per la ricostruzione e per il sostegno alla popolazione civile. Una missione politica, quindi, come ha sottolineato il ministro D'Alema, che si accompagna ad una azione diplomatica. Azioni entrambe tese ad ottenere un obiettivo strategico: aumentare la sicurezza sul piano internazionale in un'area cruciale e rilevante anche e soprattutto per tutelare la sicurezza del nostro Paese. Pertanto, lo strumento della cooperazione multilaterale e bilaterale con un impegno dell'Italia che, oltre ad un contributo straordinario, si va a sommare a risorse ordinarie, per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro circa, mi sembra il modo migliore di rimettere in moto il processo di pace, di ridurre i rischi di un sostegno di una base di massa al terrorismo, di restituire alle popolazioni di quella regione del mondo la speranza nelle istituzioni internazionali, nella logica del negoziato, nella pace. Non si può prescindere dalle ragioni dell'altro, soprattutto perché ciò permette di isolare chi ha manipolato e distorto l'immaginario collettivo della popolazione islamica, facendo leva sul contrasto tra Occidente ed Islam, sulla diffusa percezione di ingiustizia contro i musulmani per giustificare il terrorismo anche contro Stati di religione e cultura islamica moderata. La cooperazione rafforza e riempie di contenuti concreti le strategie politiche del nuovo multilateralismo, permette azioni tangibili per aiutare il popolo libanese a rafforzare le proprie istituzioni, per alimentare la volontà di dialogo, per implementare uno sviluppo di grande qualità umana e per rispondere alla necessità di allargare i contatti con l'Unione Europea e con gli altri Paesi. La cooperazione non è neutra, deve scegliere i suoi obiettivi politici e i mezzi più efficaci che ne permettano la realizzazione. L'utilizzo dello strumento militare si inserisce in questa logica di voler ricostruire le condizioni perché prevalga il negoziato, il consenso, la parola, proprio lì dove fino ad oggi hanno prevalso le armi. Questo dopo aver sperimentato, e non certo senza costi pesanti, sia sul piano della sicurezza sia sul piano delle perdite di vite umane italiane, irachene ed americane, la via della guerra unilaterale e l'illusione che la democrazia "esportata" avrebbe provocato il crollo della dittatura e diffuso pace, serenità ed altro. il fallimento in Iraq, l'inefficacia dell'intervento preventivo, oramai ritenuto tale anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, non solo dall'opinione pubblica, ma anche dai vertici militari, ci ha purtroppo dolorosamente insegnato che forse quella visione di rapporti internazionali non produce effetti positivi. Ritornano protagonisti gli organismi multilaterali (ONU, Unione Europea e NATO) e l'Italia, che all'interno di queste organizzazioni internazionali torna a giocare un suo ruolo in condizioni di parità e non di subalternità, e tutto questo nel pieno rispetto della previsione costituzionale. La differenza infatti sta tutta qui, nel multilateralismo, nella presenza dell'ONU, non certo nell'impegno delle nostre Forze armate e dell'*intelligence* che ha operato ed opera nelle missioni internazionali a fini di prevenzione dei rischi e di tutela dei contingenti militari. È giusto accogliere gli inviti giunti da più parti, *in* *primis* dal relatore Polito, a non cedere oggi, che si discute e si vota la missione Libano sostenuta da un'ampia copertura di legittimità internazionale e richiesta da entrambe le parti in contesa (Libano e Israele), a valutazioni politiche retroattive su iniziative internazionali in fase conclusiva. E' necessario, pertanto, che queste posizioni lascino ora il passo ad una più compiuta riflessione sull'esigenza di assicurare il pieno sostegno di tutte le forze politiche al disegno di legge di conversione.

Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite rappresenta una grande opportunità, ma contiene molti pericoli. Essa è nata in ritardo, dopo sei settimane di guerra e la completa distruzione delle infrastrutture del Libano e dopo oltre mille morti e migliaia di feriti, molti dei quali mutilati nel corpo e nell'anima per tutta la vita. Anche Israele ha dovuto lamentare perdite gravi e molto dolore. L'ONU insiste per garantire la pace, questa è la sua missione basica. Ma bloccare questo conflitto non è stato possibile per l'ossessione dell'ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, John Bolton, nel porre il veto al Consiglio di Sicurezza e per la pertinacia del segretario di Stato Condoleeza Rice nell'allungare i tempi, attendendo e auspicando una impossibile vittoria militare di Israele. Tuttavia, la resistenza dell'intero popolo libanese in modo unitario, l'opposizione contro l'aggressione che si è diffusa in tutti gli angoli del pianeta (in cui bisogna ricordare e collocare, come minoritaria ma esistente ed importante, quella dei pacifisti israeliani) sono riusciti a paralizzare la macchina di guerra. Ciò ha reso possibile che la diplomazia internazionale, principalmente quella europea che sui problemi della regione viveva in stato catatonico, si muovesse e desse il suo contributo alla costruzione della citata risoluzione. L'Italia ha svolto un ruolo di distacco e positivo. Le truppe con il casco blu delle Nazioni Unite, sebbene con eccessiva lentezza, si stanno schierando nel Sud del Libano. Esse dispongono di una potenza tecnologica che consente loro di rispondere ad attacchi da qualsiasi parte provengano. È questa una necessità imprescindibile perché si possa avere una separazione fra i contendenti e perché non avvenga come in passato, e anche nell'ultima guerra, in cui i militari dell'UNIFIL sono stati bersaglio di attacchi da parte delle forze armate israeliane. Riaffermiamo che il compito del contingente è di contenimento e che essi non devono mischiarsi in faccende interne degli Stati di quell'area. Notizie di un aumento dell'attività bellica ci giungono praticamente ogni ora dai martoriati paesi dell'Iraq e dell'Afghanistan. A qualsiasi persona di buon senso e di buona volontà è sempre più chiaro che le truppe straniere devono ritirarsi da quei teatri di guerra e che uno sforzo colossale va compiuto dalla diplomazia perché, dalle acque orientali del Mediterraneo alle aspre montagne dell'Afghanistan, possa germogliare il difficile e bel fiore della pace. Una volta di più, l'Europa può essere decisiva, purché abbandoni la sua assurda e autolesionista subalternità all'amministrazione di George Bush Ecco dove si presenta la sua maggiore possibilità, nel volgere la sua attenzione a quel fuoco in cui tutto iniziò e che continua ad essere la ferita aperta che contamina quell'immenso spazio geografico e complesso mosaico di popoli: la mancanza di uno Stato per il popolo della Palestina. È assolutamente inammissibile che perduri la situazione vergognosa e carica di pericoli nella quale centinaia di migliaia di palestinesi continuano a sopravvivere in campi di rifugiati, mentre tre milioni e mezzo di persone si accalcano, come in un'immensa prigione, a Gaza e in Cisgiordania: dove soffrono una situazione di carestia, di mancanza di energia elettrica, di scarsezza grave di acqua, in un territorio minuscolo che diminuisce ogni giorno, mentre assistono alla distruzione della loro cultura con le loro scuole paralizzate. Dove i Ministri sono sequestrati, le case rase al suolo da armi sempre più crudeli e sofisticate. Il numero impressionante di 750.000 palestinesi indica coloro che in qualche momento della loro vita sono già stati detenuti dalle forze militari o dalla polizia di Israele. Alcuni giorni fa in quest'Aula vi è stato un acceso dibattito intorno al discorso del Papa Benedetto XVI in Baviera. Molti onorevoli colleghi, in interventi di elevato impianto culturale, hanno difeso la figura del Pontefice e i valori del Cristianesimo. A loro, ma in realtà a tutti, desidero ricordare stralci del documento firmato dai responsabili delle Chiese cristiane di Gerusalemme l'8 luglio 2006: «La nostra sofferenza - sia palestinese sia israeliana - avrà termine quando la verità di ciascuno verrà riconosciuta. Deve essere riconosciuto il diritto di Israele di vivere in sicurezza. Allo stesso tempo però deve essere riconosciuto che il cuore del conflitto tra israeliani e palestinesi trova origine dalla privazione di libertà subita dalla popolazione palestinese (...). È contro la legge e la ragione continuare a seguire la via della morte. L'imperativo morale è chiaro. Basta con ogni tipo di violenza. Proteggere la vita e la dignità delle persone. Dare il via ai negoziati. Rompere la catena assassina di violenza dalla quale siamo tutti avviluppati Le truppe dell'ONU spiegate nel Sud del Libano non potranno, né dovranno, rimanere lì per decine di anni: questo è impossibile per motivi economici, ma soprattutto per ragioni politiche. Di conseguenza, questa missione deve essere vista solo come il primo passo di un obiettivo più ampio e complessivo: che l'Europa, e spero l'Italia, sia l'avanguardia, che incalzi i contendenti, e soprattutto Israele, per promuovere il processo di costruzione della pace e che esso possa compiere passi rapidi ed efficaci. *(Applausi dai

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, l'aggressione israeliana al Libano è iniziata il 12 luglio. Il 15 luglio, a conclusione dell'assemblea contro la guerra afghana, promossa dall'Intergruppo dei parlamentari contro la guerra, fu votato un documento conclusivo che chiedeva l'intervento dell'ONU per farla cessare. È quindi evidente che le riserve e le preoccupazioni pacifiste non vengono da motivazioni di principio ma da come la questione si è poi evoluta. Il Governo italiano ha giustamente ed opportunamente operato per un cessate il fuoco immediato e per l'invio di una forza di interposizione (anche se definire «reazione sproporzionata» una carneficina o coniare il nuovo termine di «equivicinanza» tra aggressori ed aggrediti ha creato un certo sconcerto nel movimento contro la guerra). L'iniziativa del nostro Governo ha subito trovato forti resistenze da parte di Israele e degli Stati Uniti, questo è stato sotto gli occhi di tutto e resteranno tristemente famose le affermazioni di uomini di Stato americani a fine di luglio, quando i *media* pubblicavano quotidiane notizie ed immagini di bombardamenti, di intere cittadine distrutte e di centinaia di corpi estratti dalla macerie: «Bisogna lasciare ad Israele il tempo necessario per finire il lavoro». L'Italia ha fatto bene a tentare di dare un forte ruolo di pace all'Europa ed all'ONU (in quei giorni ci fu la Conferenza di Roma ed il Presidente dell'ONU era nel nostro Paese), ma la risoluzione approvata dall'ONU, pur mettendo in conto i veti incrociati e le pressioni statunitensi, non è certo adeguata e contiene pericolose incertezze ed ambiguità. Per questo risultano poco comprensibili gli inni alla gioia che si sono, sin qui, letti e sentiti. Come si può assumere quella deliberazione sull'aggressione al Libano senza ribadire i diritti dei palestinesi ad un loro Stato, quando in Libano ci sono oltre 400.000 profughi palestinesi; senza porre il tema del ritiro di Israele dai territori palestinesi, dal Golan siriano e dalle fattorie libanesi di Shebaa; ponendo il problema del rilascio dei due soldati israeliani prigionieri in Libano senza nemmeno sfiorare quello delle centinaia di libanesi e palestinesi nelle carceri israeliane; collocando per la prima volta le truppe ONU di interposizione solo dentro i confini del Paese aggredito, il Libano? Si è quindi fermata una guerra di aggressione, ma non si sono poste le basi per modificare la situazione che l'ha prodotta. Per questo permangono forti elementi di preoccupazione. Lo stesso Presidente del Consiglio l'ha manifestata. C'è il rischio che Israele e gli Stati Uniti tornino a far salire la tensione verso l'Iran e che questo Paese si senta il prossimo bersaglio della guerra continua americana; cosa produrrebbe questo nei comportamenti delle milizie sciite, filopalestinesi e filoiraniane degli Hezbollah di fronte ad un riproporsi del tema di un loro disarmo? I nostri Governi, in Italia ed in Europa, insistono nel dichiarare che il disarmo degli Hezbollah non è un compito della missione UNIFIL, altri dicono il contrario. I giornali francesi hanno scritto che esisterebbe una stesura riservata delle regole d'ingaggio. Sarebbe quindi bene saperne di più, se non vogliamo improvvisamente trovarci tra due fuochi, in mezzo ad un teatro di guerra. E allora dobbiamo urgentemente far uscire la sinistra e tutto il popolo pacifista dalle secche dei commenti e delle posizioni tattico diplomatiche, utili forse (ma ne ho i miei dubbi) per le conversazioni di un ambasciatore e finanche di un Ministro, ma, come dimostra il riflusso del movimento pacifista italiano, letali per la chiarezza politica. È opportuno analizzare ciò che può aver spinto l'imperialismo americano sulla pericolosissima strada ora imboccata: per non rispondere del debito infinito dello Stato (50.000 miliardi dollari)? Perché nell'economia e nelle biorisorse della terra, come dicono i pensatori americani, due o più Americhe non ci stanno? Quale ne sia la causa, o l'insieme di cause, resta il fatto che siamo dentro ad una guerra continua, voluta da chi governa gli Stati Uniti per conto delle grandi *corporations* e che sta travolgendo culture, economie e diritti, in ogni parte del mondo, Stati Uniti compresi. O la fermiamo o ne saremo coinvolti e travolti. Ne discende che noi della sinistra, nonostante le divisioni, e forse in tal modo ritrovando le ragioni dell'unità, dobbiamo urgentemente aggiornare le nostre conoscenze e definire concreti obiettivi per il nostro impegno. è il momento che i segretari dei partiti della sinistra, insieme a tutti i movimenti e le associazioni contro la guerra, si facciano promotori di una grande manifestazione nazionale per l'uscita dalla guerra afghana e per scongiurare il precipitare della situazione mediorientale. Io mi impegnerò, con le mie poche forze, ad aiutare coloro che a sinistra vorranno davvero lavorare per riaprire la lotta contro questa guerra continua che è in atto e che decide e deciderà della mia vita, di quella dei miei cari e delle sorti del mondo. Ci hanno raccontato bugie colossali, e non solo sulle inesistenti armi di distruzione di massa irachene; ora dalla stampa americana apprendiamo: che il rapporto ufficiale del Governo americano su quanto accaduto il fatidico 11 settembre non regge a nessuna documentata contestazione; contestazione; che Bin Laden non è mai stato imputato per l'11 settembre, ma per aver «unicamente» organizzato attentati dinamitardi ad ambasciate americane in Africa! Noi siamo quindi in Afghanistan ed in Iraq, in guerra, uccidiamo e siamo uccisi per l'utilizzo menzognero che gli Stati Uniti hanno fatto dell'articolo 5 della Carta dell'ONU, dopo aver fabbricato un'inesistente teoria, Bin Laden-Afghanistan per farne il *casus* *belli* di una svolta che gli strateghi del Pentagono preparavano da anni. Io ho votato la fiducia al Governo sul decreto che conteneva anche la nostra partecipazione alla guerra afghana, ma l'ho fatto solo per disciplina di partito. Debbo però dare atto al Governo di avere, almeno al Senato, ascoltato le argomentazioni del gruppo di parlamentari contro la guerra e di averle ritenute lecite e rappresentative dei sentimenti e delle idee di una parte degli elettori dell'Unione; così come debbo dare atto al segretario dei Verdi, Pecoraro Scanio, di avere civilmente e democraticamente gestito i rapporti interni con i suoi senatori «dissidenti» dalla guerra. Tuttavia, superato con il voto di fiducia lo psicodramma «non fate cadere Prodi, non fate cadere Prodi», il problema c'è ancora tutto e si è aggravato: c'era l'impegno di portare in discussione tra gli stati d'Europa una chiara posizione politica del nostro Governo per l'uscita dalla guerra; nessuno ne parla più! C'era l'impegno a ridurre il numero dei nostri soldati; e si legge ovunque che sono invece aumentati. C'era l'impegno di rompere ogni legame tra la missione militare europea e quella americana di *«Enduring* *Freedom»*; leggiamo, invece, che gli Stati Uniti hanno mandato un generale a quattro stelle per dirigere tutte le forze armate operanti in Afghanistan. C'era l'impegno che i nostri militari non avrebbero preso parte alle operazioni militari decise dagli Stati Uniti per rioccupare il Sud e le altre zone che si stavano liberando dalla occupazione straniera; ora i comandi NATO ci dicono invece che tutti devono parteciparvi e che non sarebbe possibile fare altrimenti visto che lì, ora, è un inferno peggiore che in Iraq. Quando, verso fine anno, voteremo nuovamente la missione di guerra in Afghanistan, fiducia o non fiducia, io non la voterò. Non ci sono più alibi o campagne mediatiche che possano nascondere l'inganno con cui ci hanno portato, e vogliono mantenerci, in quella sporca guerra. Fernando *(IU-Verdi-Com)*. La questione palestinese è la riprova delle ipocrisie e del trionfo della politica di potenza rispetto al diritto internazionale. Io voterò a favore della conversione in legge del decreto, ma tutti: parlamentari, forze politiche, movimenti e singoli cittadini dobbiamo avere la consapevolezza che, rispetto a quello che volevamo, abbiamo ottenuto un compromesso al ribasso

a titolo personale e in dissenso dalle posizioni del mio Gruppo. Al momento del voto dichiarerò

ovvia. Ci sono elementi senz'altro positivi in questa missione, non me li nascondo. Il più positivo, e forse l'unico realmente concreto, consiste nel fatto che essa finora ha consentito una tregua. Io la considero fragile: tuttavia, è una tregua. Da quando l'UNIFIL è in

e non si raggiunge mai una soluzione. Parlo non dei poveri morti israeliani o dei poveri morti libanesi (sono tutti poveri morti, povere vittime), ma di coloro che dall'Europa o dall'America sono arrivati su quella frontiera per cercare di

Più di 50 parà francesi fecero la stessa fine: macellati con le autobombe. La missione UNIFIL 1, che è tuttora in corso, cominciò nel 1978 e quindi ha 28 anni. È una missione molto più anziana

(parlo della mia parte politica, so benissimo che questa opinione non è condivisa dalla parte opposta, o almeno da un'ampia parte dell'attuale maggioranza; ma come potremmo come potremmo noi essere più filoamericani degli americani o più filoisraeliani degli israeliani?). È bastato vedere che cosa sta succedendo per capire che la risoluzione 1701, 1701, che doveva originariamente disarmare Hezbollah - disarmare Hezbollah e basta - o provvedere affinché finalmente Hezbollah fosse disarmato dall'esercito libanese...

*(Richiami del Presidente).* Chiudo, signor Presidente, ricordando che non siamo in quei luoghi come forza di interposizione, come costantemente si dice, ma come forza che doveva garantire la fine del lancio dei missili che finora sono più di 20.000 nello stoccaggio di Hezbollah. Non esiste una frontiera fra Libano e Siria, non esiste alcun controllo su quello che succede tra Siria e Iran. Se queste sono le premesse della missione al nostro esame, purtroppo dobbiamo pensare ad un epilogo assolutamente rovinoso. La ringrazio, signor Presidente, anche per il tempo in più che mi ha concesso.

Tale novità consente per la prima volta, in quel quadrante così complicato, di far precedere una decisione politica a un intervento militare. parlare di un intervento militare; piantiamola con questa ipocrisia delle missioni di pace e delle guerre travestite da altro. Penso che usare un linguaggio razionalmente corretto sia meglio che usare il famoso linguaggio politicamente corretto,

a ragioni di partito o di parte, ma semplicemente a San Tommaso, che raccomandava a tutti di distinguere frequentemente. C'è una novità, appunto, nella questione libanese ed è una novità difficile, fragile (conosciamo tutti gli aggettivi che sono stati usati, mi associo e ne aggiungo altri dello stesso peso) e per questa ragione tengo particolarmente a che nel parlare mettiamo il luce gli aspetti di novità, non quelli di permanenza dei vecchi rischi e pericoli, perché a quel riguardo sappiamo già tutto: che le guerre fanno male lo sapeva già Omero, per dire; non è una novità particolarmente significativa.

per sostenere questo, perché bisogna proprio insistere e puntare la nostra attenzione su questi aspetti di novità politica, seguendone progressivamente i piccoli passi in avanti. La tregua dura, resiste; l'esercito israeliano si è ritirato fino al suo confine; si apre la trattativa sui prigionieri. In proposito, vorrei raccomandare che si allarghi tale trattativa, perché nelle carceri israeliane sono

del diritto, una capacità del diritto di presiedere, di governare e in qualche modo di contenere le più sfrenate passioni umane che invece non appartiene alle armi che, al contrario, stimolano gli istinti aggressivi. Non per niente gli antichi romani

questa mi pare la strada difficile che dobbiamo percorrere, quasi non ce ne sono altre. Affermo questo contro la mia consolidata opinione che non ci sia mai una soluzione sola per un qualsiasi problema. Tuttavia, qualche volta si pongono necessità così pressanti

associarmi al voto che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha deciso di esprimere, vale a dire l'assenso a questa missione. Non lo so e quindi in questo senso, pur esprimendo con la massima sincerità il mio pensiero, il mio resta un intervento personale.

difficile e onerosa»; di questi tre aggettivi sicuramente quello che resta vero è che sarà non onerosa, ma onerosissima:

Se, per esempio, si apprende che dall'Iran o da un porto della Siria parte una nave che contiene armi armi potenti o che, comunque, possono colpire Israele e questa, sempre attraverso un'informazione che sia precisa, si sa che non è stata fermata e non è stata nemmeno controllata dalle navi libanesi, che cosa può e deve fare la missione Leonte e, in questo caso in modo particolare, la missione affidata alla nostra marina? Potrei continuare a lungo su questa strada. Ecco la ragione per la quale, onorevole Forcieri, ormai davvero considero questa missione con una denominazione che sarebbe singolarissima:

ed infine per indurre l'Iran a mettere fine alle minacce di distruzione di Israele. Se, però, di fronte ai casi specifici che ho indicato e per i quali attendo una risposta dal Governo, non vi è una possibilità operativa e militare,

a questa missione militare di pace, in cui l'Italia impiega il massimo di potenzialità militare,

e con l'iniziativa prevista dalla risoluzione 1701 ha ampliato il mandato della precedente missione UNIFIL con un vasto protagonismo europeo, consentendo, con il consenso delle parti (elemento fondamentale), il cessate il fuoco e la tregua. tregua. Voglio ricordare che lo scenario politico dell'area è comunque allarmante e legato ad equilibri complicati e precari. Non vi è dubbio che le dubbio che le guerre preventive dell'amministrazione Bush, invece di risolvere il problema del terrorismo, hanno agito da detonatore ampliandolo. comunque che il mantenimento della tregua tra Libano e Israele e la costruzione politica della pace e la stabilizzazione del Libano

Palestina-Israele) e dagli autori indiretti, come li chiama Caracciolo, gli «*sponsor»* (gli Stati Uniti e l'Iran), che hanno diversi interessi geopolitici che li distinguono. Nell'area si giocano diverse partite di grande importanza per la stabilità dell'intera regione: quella ideologico-religiosa, che concerne non solo la questione «fondamentalismo contro Occidente», ma anche lo scontro religioso e politico religioso e politico fortissimo tra sciiti e sunniti, che vediamo dispiegato in Iraq anche in questi giorni. Inoltre, la partita energetica (i gasdotti afgani, il petrolio iracheno, il recentissimo oleodotto BTC, che collega il Mar Caspio al porto turco di Ceyhat), partita che, da parte degli Stati Uniti, mira ad isolare l'Iran e a rendere le sue riserve energetiche sempre meno strategiche per il mercato mondiale. L'Iran, a sua volta, vuole sottrarre il mercato petrolifero al dollaro per passarlo all'euro. Un'ulteriore partita è quella che riguarda il nucleare iraniano ed è partita delicatissima, con conseguenze dirette sulla stabilizzazione del Libano. È come dire che l'Iran accetta di buon grado questa missione - controllando che Hezbollah non l'ostacoli se l'Iran stesso verrà coinvolto nella stabilizzazione dell'area, se non sarà a sua volta attaccato e non verrà messo in discussione il suo Governo e, se infine, sul nucleare si procederà ad una trattativa diplomatica e politica che deve continuare. Che l'Iran utilizzi l'uranio per fini civili è un suo diritto. Dovranno esserci i controlli e le ispezioni dell'AIEA; e questa è una via, però, se le ricerche e le sperimentazioni dell'Iran mirano alla costruzione di armi atomiche, è chiaro che ciò costituisce un ulteriore elemento di instabilità e di rischio. Ma le spinte dell'Europa e del resto del mondo per un Medio Oriente denuclearizzato dovrebbero valere per tutti, a cominciare dalle 200 testate nucleari già a disposizione di Israele. Non solo: le ragioni per impedire all'Iran di avere l'atomica diventerebbero cogenti se, su scala mondiale, venisse rilanciata la proposta del disarmo chimico, batteriologico e nucleare. Chiediamo allora al nostro Governo di farsi promotore nelle sedi internazionali di una conferenza regionale che coinvolga tutti i Paesi dell'area in cui, oltre alla ricerca di percorsi per prevenire i conflitti e di stabilizzazione della pace, sia prevista anche la denuclearizzazione

incidenti anche non premeditati possono mettere in discussione, inducendo una spirale dagli esiti incontrollabili. Molti analisti, poi, "gufano" un po' e parlano di questa tregua come di una pausa che può preludere a scenari di conflitti dirompenti;

è riesploso il dibattito sulle regole di ingaggio della missione, di cui abbiamo molto parlato, Sottosegretario, anche in Commissione, riportate dal quotidiano spagnolo «El Pais». Pais». Fino dalla fine di agosto si era detto che il mandato ONU le prevedeva «robuste»: i francesi, memori - lo ricordava il collega Guzzanti prima - dei 58 paracadutisti uccisi nel 1983 da una autobomba, avevano preteso l'uso della forza preventiva non solo in caso di possibili attacchi, ma anche per impedire Ma quali attività sono ostili? che parlava di assistere l'esercito libanese perché disarmasse Hezbollah. Ricordo le parole del generale Castagnetti, molto autorevole, a cui tra l'altro va il merito il merito - e lo sottolineo - di avere operato per l'efficacia della catena di comando, ottenendo la costituzione all'ONU di un'apposita cellula strategica per dirigere la missione. Ricordo che questa cellula strategica è fondamentale per non incappare negli stessi errori in cui si era incappati a suo tempo in Somalia. Il generale Castagnetti dice, a proposito delle regole di ingaggio, che se si incontra un camion di armi di Hezbollah, visto che non si ha il compito di disarmarlo, ma di assistere le forze libanesi, il buon senso lo porta a pensare che il compito sarà quello di avvertire l'esercito libanese affinché il camion venga

l'UNIFIL dovrebbe operare nell'assistenza alla popolazione civile, all'esercito libanese e come interposizione. A quanto dice «El Pais», le regole d'ingaggio ampliano lo spettro di azione e la non belligeranza con Hezbollah potrebbe essere a rischio, dal momento che UNIFIL metterà posti di blocco sulle strade libanesi e, come si legge, procederà direttamente al sequestro delle armi se l'esercito libanese non è in grado di farlo. farlo. Il quadro è allarmante, anche se fino ad oggi - leggo evidentemente giornali diversi da quelli del collega Selva - pare che le violazioni della tregua (a detta del portavoce di UNIFIL, Alexander da parte di Hezbollah sono state vicine allo zero, contro le oltre cento da parte israeliana, senza contare le violazioni dello spazio aereo libanese. Mi preme segnalare un ultimo punto, Presidente, che ha agitato molto il dibattito nelle ultime settimane; ne abbiamo parlato anche in Commissione difesa. L'articolo 188 della finanziaria, che prevede il finanziamento triennale delle missioni, prevede appunto che il finanziamento venga autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio, per le missioni deliberate dal Consiglio dei ministri. ministri. Dietro questa formula, in realtà, assistiamo ad uno scippo al Parlamento del potere decisionale; resta solo un generico atto di indirizzo da parte del Parlamento per il quale non sono specificate né la portata, né l'estensione, né la validità. validità. Non solo: il terzo comma stabilisce che tale previsione si applica anche al finanziamento delle missioni in atto. Signor Presidente, le missioni all'estero sono la principale attività di politica estera e di difesa del nostro Paese; ne lamentiamo da tempo lo schiacciamento del dibattito e delle decisioni alla sola scadenza del finanziamento, ma ma abolire anche questo residuo di confronto e di decisione parlamentare significa andare in direzione opposta, esautorando il Parlamento da una sua irrinunciabile prerogativa.

vorrei effettuare alcune considerazioni, ponendo alcuni interrogativi. È chiaro che ai nostri militari impegnati in Medio Oriente vanno tutto il mio personale sostegno e tutta la mia stima per il servizio che sono chiamati a rendere alla comunità internazionale; questa missione, però, non poche incongruenze, sia sul fronte interno sia su quello internazionale. È una partita al buio, quella che si sta giocando in Libano, anche se sotto l'egida dell'ONU: tutti gli interrogativi posti sulle regole di ingaggio ad oggi sono rimasti inevasi e, com'è noto, è da queste regole che dipende la possibilità, per i nostri soldati, di fare ricorso alle armi per difesa. L'elasticità nei comportamenti lasciata ai nostri militari in caso di minaccia rappresenta, di per sé, una pericolosa in un'area in cui la politica sposa l'estremismo religioso, più fedele all'uso del *kalashnikov* che alle regole del Corano. È un aspetto tutt'altro che marginale, nella regione più calda del Libano, ancora in mano alle milizie di Hezbollah, un movimento che, in questi giorni di un dopoguerra instabile, ha trovato il modo, il tempo il tempo e gli spazi per celebrare in piazza quella che ritiene una vittoria ai danni d'Israele. Ma poi, chi sorveglierà la frontiera con la Siria, che nei mesi scorsi ha rifornito di armi gli estremisti islamici? Giusto alcune settimane fa, il *leader* del partito di Dio Nasrallah ha dichiarato che nessun esercito al mondo potrà disarmare Hezbollah ed ha dato il benvenuto alla forza multilaterale UNIFIL, ma a condizione che non spii la resistenza e non tenti di disarmarle la resistenza, né interferisca negli affari libanesi. Sono parole inquietanti, che spiegano come questi terroristi - perché di questi si tratta - abbiano ancora un controllo significativo sul territorio e sul tessuto socio-politico libanese. aspetti tutt'altro che marginali, per le conseguenze che potrebbero avere sulla sicurezza dei nostri soldati. Occorre, poi, valutare le conseguenze politiche della missione in Libano: dal Governo e dalle forze di maggioranza giungono appelli al voto *bipartisan* in nome di una sorta di responsabilità politica che dicono essere comune, di fronte all'ONU ed al mondo intero, che guarda con apprensione a quel che accade - com'è giusto che sia - fra Israele, Libano e Palestina. E che dire del fatto che il Governo aveva dichiarato che la missione sarebbe partita solo ove avesse ricevuto il sostegno del Parlamento? I nostri soldati, in realtà, sono già là, senza e prima ancora di aver ricevuto il sostegno parlamentare. Il Governo aveva concordato che la missione sarebbe stata inserita nella politica europea, nel senso che doveva ricevere l'adesione ed il concorso di venticinque Paesi europei: ma, in realtà, l'Italia ha offerto il 40

aveva indicato il generale Castagnetti come capo della missione, ma questi è stato sostituito perché non godeva del gradimento di Kofi Annan. Anche tale inaccettabile imposizione al Governo italiano, però, è passata irrimediabilmente sotto silenzio. Non possiamo, poi, dimenticare che coloro che oggi invitano la Casa delle Libertà ad appoggiare la missione in Libano sono gli stessi che, fino a qualche mese fa, avevano apertamente ostacolato l'invio di militari in Iraq. Dunque, mi chiedo: dove sono i pacifisti di allora? Dove sono finite le migliaia di bandiere della pace che sventolavano dai balconi e ad ogni comizio? Sono diventati tutti militaristi? Quelle bandiere non si vedono più: sono state ammainate, perché, forse, vi sono missioni di pace più giuste di altre? Oppure, oggi, come in Iraq e come in Afghanistan, l'Italia è chiamata a difendere i valori della democrazia e della libertà, che non conoscono distinzioni di sorta? Ora che i nostri militari sono tornati dal martoriato Iraq, non vorrei che ci si dimenticasse in fretta del servizio che hanno prestato per anni, a volte pagando con la loro vita. Non credo che la maggioranza e il Governo possano nascondere dietro l'invito fatto all'opposizione ad una collaborazione sulla missione in Libano le loro incongruenze e le loro lacerazioni interne. Non credo che questo Governo possa pensare che allargando il numero dei voti parlamentari, da un lato, aumenti il peso politico di una scelta e, dall'altro, vada a dissipare le perplessità del centro-sinistra. È tempo che questo Governo e questa classe politica si assumano le loro responsabilità di fronte agli elettori. È tempo che questo Governo, in mancanza di numeri, non cerchi legittimazioni esterne, comodi salvagenti per le sue decisioni. Ecco perché, a mio parere, dovrebbero approvare la missione in Libano contando solo sui loro voti, senza contare sulla sponda di comodo tra i banchi dell'opposizione. Per questo il mio voto potrebbe essere aggiuntivo - starò a vedere quello che succede ma mai sostitutivo di quello della maggioranza. Abbia questo Governo il coraggio di difendere fino in fondo le proprie scelte di fronte all'opinione pubblica e di fronte agli elettori. Ne guadagnerebbero il senso di responsabilità, la coerenza, il rispetto della gente.

del Governo nelle sue massime espressioni, ma anche di quasi tutti i colleghi senatori, magari quegli stessi che soltanto otto mesi fa, dietro striscioni pacifisti, su temi pacifisti come questi, manifestavano per la pace e la libertà e contro il Governo Berlusconi; magari gli stessi che avrebbero gremito quest'Aula qualora questo argomento fosse stato trattato soltanto otto mesi fa per dire che questa missione «non s'ha da fare». Oggi, evidentemente, sono impegnati in qualche corteo della stessa natura. È con tristezza che sottolineo le assenze del Governo e del Ministro della difesa, rispettando le presenze che al contrario ci sono, ma che comunque non sostituiscono coloro i quali debbono poi prendere le decisioni e rappresentare il Paese riguardo a quelle stesse decisioni. Mi spiace anche sentire

Cara senatrice, è la nostra stessa preoccupazione perché voi non siete né coesi, né uniti e non siete d'accordo su temi che coinvolgono l'interesse del Paese.

prima di esprimere il nostro parere sull'attuale missione, che vede coinvolte le truppe italiane in Libano, non possiamo non riportare alla memoria dei presenti e di tutti i cittadini le prime due missioni, di cui si è tanto parlato durante il Governo Berlusconi, aspramente criticate e portate come vessillo di una sciocca guerra contro il precedente Governo. A consuntivo, si sono rivelate a dir poco utilissime ai fini del perseguimento della pace e dello sviluppo di quei martoriati luoghi. I nostri caduti sono considerati unanimemente e a tutti gli effetti eroi della e per la pace. La loro memoria e il loro sacrificio esigono rispetto assoluto. È inoltre doveroso riconoscere come i soldati italiani non abbiano sparato un colpo, mentre i medici presenti nelle truppe hanno effettuato migliaia di operazioni e portato aiuto, distribuendo medicinali e soccorso senza mai risparmiarsi. Sicuramente si è trattato di missioni caratterizzate da una presenza fisica volta per lo più all'organizzazione e alla distribuzione delle risorse necessarie e indispensabili per la sopravvivenza di larghe fasce della popolazione locale. Le fasce più deboli della società afghana, ad esempio, hanno mostrato più volte di apprezzare, anzi, di richiedere con insistenza la presenza dei nostri soldati, visti come una speranza per il miglioramento delle tristi condizioni di vita in cui giacciono i loro figli. Chi invoca a gran voce il ritiro e il ritorno in Patria dei nostri soldati da quei tristi luoghi, martoriati da anni di guerra, si professa falsamente progressista, poiché è troppo semplice far finta di ignorare cosa ciò comporterebbe in quei Paesi.

in segno di continuità con le scelte effettuate durante la precedente legislatura ed in ossequio all'articolo 11 della nostra Carta costituzionale. Non possiamo fare a meno di ricordare come le prime missioni, dichiaratamente di pace, siano state aspramente criticate in molte piazze come missioni di guerra e portate come vessilli di una opposizione al Governo Berlusconi. La missione in Libano, per la quale noi voteremo, a causa della posizione geografica di quel Paese, del fatto che risulti sotto l'influenza Hezbollah, attaccato per tale motivo da Israele sino a poco più di due settimane fa e tenuto sotto stretta vigilanza dalla Siria, è rischiosa per le è rischiosa per le nostre truppe, anzi, forse è la più rischiosa tra le missioni sinora partite. Inoltre, non possiamo, trascurare la forte incidenza che essa sul piano finanziario per il nostro Paese, sottoposto proprio in questi giorni alle continue minacce di una finanziaria oppressiva ed onerosa. Certo, non cambieremo la nostra opinione rispetto alle scelte già effettuate a suo tempo, ma siamo sicuramente sconcertati dal comportamento degli esponenti di questo Governo che in precedenza ci hanno accusato di essere dei guerrafondai mentre ora si rivestono dei panni dei portatori di pace, grazie anche all'ausilio di cui godono da parte di alcuni *media*. Speriamo che questa missione non si trasformi in uno *slogan* meramente promozionale del Governo Prodi e della comunità internazionale in un periodo così difficile come quello dell'approvazione della finanziaria, ove da più parti si raccolgono i malumori del popolo italiano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono d'accordo. Vorrei scandire queste parole perché nel momento in cui ci accingiamo ad un voto così importante ritengo opportuno, sotto l'aspetto politico e personale, che ognuno di noi, e me per prima, faccia chiarezza. Non sono d'accordo per le perplessità sulla matrice di questo decreto: restano misteriose, per doverosi motivi di sicurezza, le regole di ingaggio che rappresentano le pietre miliari dell'impegno dei nostri militari in Libano, ma non possiamo nasconderci come la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'ONU non affronti, se non in maniera sfumata, il nodo della situazione nell'area, e cioè la collaborazione del contingente UNIFIL al disarmo delle milizie Hezbollah. Una decisione che sarebbe stata coraggiosa e che però non si è voluto o potuto prendere; una decisione che avrebbe, questa sì, contribuito alla pacificazione dell'area. E allora, la risoluzione e l'impegno dell'ONU in Libano troppo da vicino ricordano precedenti risoluzioni e precedenti impegni nella ex Jugoslavia o in Africa che hanno visto i caschi blu muti ed impotenti testimoni di massacri. Quanto poi quell'ignavia abbia pesato nella considerazione delle Nazioni Unite come reale strumento di pace potete ben immaginarvelo. Le immagini di quei corpi straziati, di quelle fosse comuni, restano un'indelebile vergogna per tutte le Nazioni civili e non vorrei che nei prossimi mesi un'altra vergogna si aggiungesse a quella che già proviamo. Tuttavia, la politica, l'arte del possibile a favore della comunità, ha in mano una bilancia dove ai contro vanno contrapposti i pro, e sono questi pro a farmi al momento propendere verso un voto favorevole. Il primo: occorre che la risoluzione ONU, per quanto blanda, possa essere osservata alla lettera, senza ulteriori mitigazioni, e per questo occorre una vigilanza e un sostegno, il più possibile ampio, alla missione. Il secondo: l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati, che riconosce come missioni di pace le operazioni condotte all'estero da questo e dal precedente Governo, rappresenta un'opera di verità preziosa. Voglio sperare che quel voto, così ampio, fosse una vera presa di coscienza democratica e non dettata da tatticismi parlamentari, che poco hanno a che fare col campo delicato della politica estera. Ma sarà un voto da verificare costantemente, un'apertura di credito da parte nostra, condizionata, per evitare che la maturità, così velocemente conquistata da ampi settori del centro-sinistra,

che si rifiuta di dire "mangiatevela voi, oggi, questa minestra", che si rifiuta di piegare alla ricerca di un facile consenso le ragioni alte del nostro stare insieme, e che intende contribuire attivamente alla ricerca di una religione civile comune che possa, a prescindere dalle maggioranze che si alternano alla guida del Paese, sorreggere sempre le nostre decisioni quando siamo chiamati a scegliere tra il giusto e l'ingiusto, tra dittatura e democrazia, tra oppressione e libertà. Una *union sacrée* che dovremmo sempre ai nostri militari e che sempre la sinistra, quando si è trovata all'opposizione, ha rotto. Oggi, se le condizioni del dibattito in quest'Aula ce lo consentiranno, vorremmo invece realizzarla, sperando che, quando le parti di maggioranza e opposizione, in un tempo che ovviamente mi auguro breve, saranno invertite, il nostro esempio verrà seguito qualora, in futuro, la comunità internazionale, l'Occidente e, consentitemelo, quella parte d'Occidente e d'Europa che si chiama Israele, ci debbano chiedere un nuovo impegno per la pace, la libertà, la tutela del diritto delle genti e dei popoli. Presidente, il mio sarà un intervento a titolo personale. Francamente, su un tema così complesso e così serio ci sarebbe stato bisogno di un'analisi approfondita. Il tempo che mi è concesso non me lo permette. Farò, quindi, alcune osservazioni che mi sembrano essenziali. Per cominciare, questa è una missione formalmente pacifica, ma realisticamente è una missione che potrebbe rivelarsi più pericolosa di altre che da parte dell'attuale maggioranza sono state criticate e combattute. Tutti gli esperti militari e gli osservatori politici sono consapevoli che gli scopi prefissati di questa missione non verranno mai raggiunti che anzi essa potrebbe addirittura produrre guasti molto seri. Lo scopo è la pacificazione,

una giornalista informata e molto seria. Già il titolo dell'articolo è significativo: «La quiete prima della tempesta». Seguono notizie davvero allarmanti: armi che arrivano tuttora dalla Siria agli Hezbollah; Damasco che seguita ad ospitare e a coordinare azioni terroristiche. Questo è quanto denunciato dall'articolo della Nirenstein. L'Esecutivo libanese, l'esercito libanese, è, in pratica, connivente con gli Hezbollah, dice la Nirenstein, e l'UNIFIL, com'è detto nella risoluzione ONU, deve segnalare all'esercito libanese dove e come gli Hezbollah nascondono o esibiscono armi. Ebbene, l'esercito libanese, e questa è una denuncia davvero preoccupante, evita accortamente di intervenire e anzi avverte addirittura gli Hezbollah di allontanarsi. Queste sono denunce molto serie, molto allarmanti, sulle quali vorrei che il Governo oggi, prima del voto, fornisse dei chiarimenti. Serve a qualcosa ricordare che due risoluzioni dell'ONU sono ignorate? La 1559, per esempio, che impone il disarmo degli Hezbollah, e la 1701, che impone all'UNIFIL di collaborare con l'esercito libanese perché ristabilisca il pieno controllo dell'area. Ma c'è di peggio, e questo peggio ci riguarda direttamente: Hezbollah, tramite un suo importante dirigente, Nabil Kauk, in occasione proprio della recente visita visita dell'onorevole Prodi in Libano, dopo aver dato il benvenuto al nostro Primo Ministro, ha ammonito l'Italia perché le nostre truppe non eccedano nella pretesa di esercitare un controllo

realtà del Libano, molto più pericolosa di quel che appare dalle dichiarazioni ufficiali del nostro Governo. Mi chiedo come si è potuto gridare allo scandalo e fare tante manifestazioni e dichiarazioni per l'invio di truppe in Iraq e in Afghanistan e far passare questa missione in Libano come pacifica e senza rischi.

diciamo così, contrario a quei ragazzi che sono in Libano e fanno il loro dovere. Ma non posso votare a favore, stante questa ambiguità, che è ambiguità politica esercitata dal Governo, dalla classe politica italiana, dalla maggioranza; ambiguità militare addirittura sul posto, dove UNIFIL sopporta che l'esercito libanese non faccia controlli seri e accetta addirittura questa situazione equivoca per cui ancora dalla Siria arrivano armi agli Hezbollah e gli Hezbollah le esibiscono e minacciano. Quindi, francamente non si può dire, almeno per quanto mi riguarda, sì La mia astensione vuole essere un richiamo alla realtà del Libano, a non affidare la sorte dei nostri ragazzi, dei nostri soldati all'ambiguità agli equivoci e agli inganni di una situazione carica di rischi seri. Concludo dicendo che mi piacerebbe, il che potrebbe addirittura convincermi a votare diversamente, che il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio o almeno del Ministro della difesa, venisse in Parlamento e dicesse con chiarezza quel che accade in Libano, qual è il comportamento. Chiedo al Ministro

Signor Presidente, colleghi senatori, ieri a New York, durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

in Assemblea sono un segno importante della centralità acquisita dalla nostra politica estera in questo momento per la particolare congiuntura a livello internazionale.

sulle missioni internazionali, afferma con nettezza il ripudio da parte della Repubblica italiana della guerra come strumento di offesa e per la soluzione delle controversie internazionali.

non può esistere la pace in un solo Paese o in una sola area del mondo e chi crede nel valore fondamentale della pace deve lavorare perché essa si estenda e, soprattutto, raggiunga aree che non la vedono affermata ma, anzi, quotidianamente Questo interventismo per la pace, questo non isolazionismo, questo pacifismo non isolazionista del nostro articolo 11 ha ispirato una linea di politica estera di lungo periodo che ha contraddistinto l'intera

il principio del multilateralismo, come strumento privilegiato per un interventismo a favore della pace e della democrazia nel mondo.

Mediterraneo può diventare l'epicentro di un catastrofico conflitto mondiale oppure può, e deve, diventare luogo di alimentazione di una nuova stagione di pace e di incontro tra i popoli. Questa linea di politica estera è risultata utile in un passaggio cruciale, quello che ha portato dalla tragica guerra in Libano alla fragile tregua nella quale siamo impegnati in questo momento.

Credo che il tormento sincero che tanti colleghi del centro-destra hanno espresso questa mattina e che io rispetto, anzi, apprezzo per la linearità e per l'onestà intellettuale - vorrei dire di più - sia condiviso

il ruolo dell'Italia nel mondo e per la sua politica estera. Come ho già detto in Commissione e voglio ripeterlo in che penso non sarebbe stato saggio compiere se non ci fosse stato l'appoggio e il sostegno da parte dell'opposizione, perché ci troviamo di fronte

alberghi nell'animo di tutti i senatori e di tutti i Gruppi che fanno parte del Senato; reputo, quindi, che aver messo in luce tale difficoltà e questo tormento di coscienza da parte di di molti senatori del centro‑destra rappresenti un passaggio parlamentare importante che deve essere raccolto e rispettato. La missione è doverosa,

con l'onestà intellettuale che tutti gli riconosciamo il senatore Guzzanti - oggi saremmo ancora in presenza di un conflitto di quelle proporzioni, che probabilmente avrebbe potuto estendersi in tutto il Medio Oriente. Oggi ci troveremmo in una situazione drammatica e tragica per il Medio Oriente e, forse, per l'umanità. Ciò spiega probabilmente anche il successo della risoluzione 1701.

i contendenti e protagonisti di quel conflitto erano i primi a sapere che non potevano andare oltre un certo punto senza scatenare l'inferno. Quindi, la risoluzione 1701, per la prima volta nella storia, è riuscita a fermare un conflitto, perché come dire - eravamo sull'orlo di un abisso. Quindi, ci sono stati il coraggio e la lucidità di fermarsi e l'Italia ha dato il suo contributo: credo che sia importante rimarcarlo e sottolinearlo perché è un contributo del nostro Paese, non solo del nostro Governo. Si tratta di un apporto che il Nostro Paese ha dato fermare una guerra, consentendo quella fragile tregua rappresentata dalla risoluzione 1701. Questo è il carattere doveroso di quella missione. Essendo stati noi a sostenere che bisognava

il comando e la responsabilità di questa nuova istituzione, cioè la cellula strategica militare a New York, che è un altro passo avanti importante e significativo nel quale dobbiamo mettere alla prova la nostra capacità, professionalità e il nostro coraggio.

stabilire una forza d'interposizione che deve sostenere il Governo libanese nel disarmo di Hezbollah, deve tutelare i confini di Israele e, in qualche modo, presidiare ad una fragilissima tregua in un contesto nel quale i bacini di odio hanno una profondità e un'estensione drammatica e nel quale ci sono gli arsenali di guerra più importanti del mondo, dopo quelli delle superpotenze atomiche.

il primato della politica e della diplomazia. Il successo di questa missione militare dipende strettamente dal successo dell'iniziativa politica dei prossimi mesi e il tempo è drammaticamente breve.

per un'iniziativa politico - diplomatica a livello internazionale. Pertanto, o questa iniziativa viene assunta e l'Italia riesce anche ad utilizzare il patrimonio di credibilità

per un'iniziativa di pace e di stabilizzazione dell'intera area mediorientale o, altrimenti, è chiaro che la nostra missione è a termine e ad un termine molto breve. Infatti, qualora lo scenario dovesse degenerare è difficile immaginare un futuro per la nostra missione militare. Il senatore Selva parlava prima, con l'arguzia intellettuale che gli è propria, di una missione militare senza sparare: noi ci auguriamo che questa missione sia tale. Vorrei ricordare al senatore Selva, che in questo mi è maestro, che la più grande e gigantesca missione militare senza sparare è stata quella della NATO che ha vinto la guerra fredda senza sparare un colpo.

la ragion d'essere della nostra missione verrebbe meno, dovendo a quel punto diventare una missione schierata da una parte o dall'altra, ma certo non potrebbe farlo con i caschi blu; in caso contrario, non ci resterebbe che prendere atto del fallimento dell'iniziativa politica e del suo braccio militare.

la consapevolezza e la constatazione dell'impossibilità di arrivare ad una sistemazione e ad una stabilizzazione del Medio Oriente e a una soluzione della crisi israelo-palestinese senza coinvolgere i vicini, gli ingombranti vicini di casa: la Giordania, la Siria e l'Iran. In particolare, credo che sia indispensabile una strategia sull'Iran che in questo momento la comunità internazionale non ha: non c'è ora una vera strategia sull'Iran. È difficile È difficile averla, ma dobbiamo costruirla, perché è questo adesso il passaggio probabilmente decisivo per arrivare alla stabilizzazione dell'area Sulla questione iraniana la linea di politica estera condotta dall'amministrazione Bush in questi anni è un affollarsi di contraddizioni e paradossi. Probabilmente l'Iran, che è l'interlocutore decisivo e anche quello più pericoloso per la stabilità e la pace a livello internazionale, è stato fortemente avvantaggiato sia dalla guerra in Afghanistan, sia da quella in Iraq.

imposto attraverso sanzioni che non sono credibili e la minaccia di un intervento armato che è ancora meno credibile. So di avventurarmi su un terreno molto difficile, un crinale rischioso e scivoloso, tuttavia la strada è quella. Non possiamo pensare di affrontare

Tale suggerimento deriva anche dall'esperienza di questi giorni e di queste settimane. È necessaria una vera e propria offensiva diplomatica nei confronti dell'Iran, che in qualche modo riconosca il suo diritto alla sovranità energetica attraverso la tecnologia nucleare, ma che nello stesso tempo tempo passi attraverso il riconoscimento da parte dell'Iran stesso della sua possibilità di giocare un ruolo di stabilizzazione e di pacificazione dell'area, rassicurando i suoi vicini e la comunità internazionale. Si tratta di un percorso molto stretto,

come portatori di un'alternativa di fondo al cosiddetto unilateralismo bushista, ma vi siamo soprattutto per contrastare Israele. La nostra presenza in Libano è soprattutto diretta ad impedire che Israele si difenda dal terrorismo sciita

perché siamo contro l'unilateralismo, ma siamo equivicini sia ai terroristi di Hezbollah*,* sia ad Israele. Non siamo lì per contrastare Israele, come intende la sinistra radicale. infine, un'altra lettura di questa missione, minoritaria all'interno del Governo. Si tratta di una lettura che in un primo momento è stata offerta anche dallo stesso ministro della difesa vogliamo applicare e vogliamo che sia applicata la risoluzione 1701 dell'ONU, che prevede il disarmo delle milizie. Le risoluzioni dell'ONU, signor Presidente, sono quello che sono. La risoluzione dell'ONU 1559 del 2004 prevedeva il ritiro delle truppe siriane, la presenza dell'esercito libanese nel Sud, che doveva sostituire e neutralizzare le milizie terroristiche di Hezbollah, e lo smantellamento, quindi, di tali milizie. Quella risoluzione non ha mai trovato applicazione, se non per il ritiro dell'esercito siriano che fu provocato da eventi interni al Libano.

quella sciita a cui si rifà Hezbollah, quella drusa, quella cristiano-maronita e vi sono altre comunità cristiane che, in contraddizione con la cristiano-maronita, stanno tentando un approccio con gli sciiti di Hezbollah. in sostanza, è un crogiolo di culture, di presenze, di entità e di identità. Quindi, quando si affronta un problema come quello libanese lo si deve fare con sistemi di lettura e di intervento quanto mai sofisticati. A dire la verità, lascia interdetti la grossolanità e la ruvidezza

Il mancato successo dell'offensiva israeliana nei confronti delle milizie terroristiche di Hezbollah ha creato un nuovo scenario geopolitico in Medio Oriente ed enormi problemi agli stessi americani perché un Medio Oriente, nel quale il potere di interdizione e di deterrenza israeliano si è enormemente indebolito, è un Medio Oriente che entra in una fase di impressionante se siamo consapevoli - e se sia consapevole il Governo - che nel momento in cui accettiamo di essere presenti in Libano, in realtà, non è per contraddire Bush e l'unilateralismo bushista,

signor Presidente, dobbiamo essere consapevoli che in Libano ci siamo anche perché gli americani ci hanno voluto e hanno voluto l'Europa affinché fosse

ha solo conosciuto una delle sue fasi periodiche di trattativa)

La grande rivoluzione sciita, che sta contaminando l'Islam, è qualcosa di storicamente terribile perché produce una destabilizzazione a livello dello stesso mondo islamico: gli sciiti, signor Presidente, sono una minoranza del 15 ma anche la minoranza degli esclusi. Sono una minoranza che ricorda un po' l'eresia catara. Immaginate se all'interno del cristianesimo improvvisamente l'eresia catara, invece di essere fermata

deve sorgere o fuoriuscire da una caverna nella quale dorme. Tutto questo mondo, pari al 15 per cento dell'Islam, è in attesa millenaristica di questo dodicesimo Imam, che dovrà riscattare l'umanità e gli sciiti che, fino ad ora, erano gli esclusi del mondo islamico. Noi andiamo a porci in quella realtà e questo Governo deve essere consapevole delle sue scelte e delle conseguenze delle sue scelte. Altro, caro collega, che intervento disarmato! Ne parleremo tra qualche anno

Però sappiamo anche, per coerenza e per lealtà verso l'alleato non bushista, verso l'alleato americano e per coerenza e lealtà verso Israele, che in questo momento dobbiamo esserci, ma non contro Israele e contro gli Stati Uniti, ma con Israele e con gli Stati Uniti.

ed il contenuto di un ordine del giorno presentato da altri colleghi del Gruppo di Rifondazione comunista - Sinistra europea che, in linea di massima, raccoglie alcune delle sollecitazioni e delle osservazioni svolte anche dal collega Tonini riguardo all'urgenza di un percorso che porti ad una Conferenza internazionale di pace. Ha detto bene il collega Tonini: le questioni sono indissolubilmente intrecciate. La risoluzione 1701 ha ha vari obiettivi: il primo certamente di inviare una forza di interposizione che potesse comportare come conseguenza la cessazione delle ostilità; il secondo di assistere il Governo libanese nella messa in sicurezza del confine e dal punto di vista politico aprire gli spazi per una soluzione politica, con le armi in silenzio. Tuttavia, non possiamo noi oggi accontentarci di quel primo passo verso la giusta direzione. Gli spazi di manovra sembrano oggi estremamente ridotti. Lo stesso *International Crisis Group*, un importante centro di ricerca, proprio nei giorni scorsi, ha prodotto un *briefing* molto interessante che analizza le opportunità e le possibilità per costruire una soluzione politica, riconoscendo comunque che oggi quasi tutti gli indizi vanno contro e che, comunque sia, la situazione sul campo è estremamente delicata e richiede uno sforzo forte da parte della comunità internazionale. Quindi, è una finestra di opportunità che dobbiamo essere in grado di cogliere subito perché l'opportunità politica che ci si presenta davanti con l'entrata nel Consiglio di sicurezza è importante e può capitalizzare**,** anche con l'iniziativa politica svolta dal nostro Paese fin dall'inizio della crisi libanese, poi sfociata nella Conferenza di Roma ed in un forte impegno nella partecipazione a UNIFIL 2. Tuttavia, come ho detto, questa iniziativa non può limitarsi a ciò; non possiamo accontentarci dell'uso dello strumento militare per la soluzione delle controversie e delle crisi internazionali, anche se, in questo caso, nel quadro di un'azione multilaterale, legittimata dall'ONU, ci è sembrato un elemento importante e imprescindibile. Cosa significa oggi il nostro ordine del giorno? Significa che invitiamo il Governo a proseguire nella strada già intrapresa con una serie di colloqui importanti ad alto livello - anche la visita del Presidente del Consiglio in Libano rientra in questa ampia strategia - che di fatto riconosce un punto, ossia che il secondo passaggio previsto dopo la risoluzione 1701, ovverosia un'altra risoluzione del Consiglio di sicurezza, che doveva costruire i tasselli di una soluzione politico-diplomatica, tarda a venire. In tal modo rischia di chiudersi quella finestra di opportunità che, a nostro parere, bisogna continuare a tenere aperta, attraverso un lavoro per una Conferenza internazionale di pace, che tenga insieme tutti quanti gli elementi: il problema interno al Libano del reintegro di Hezbollah come movimento politico, e quindi il suo disarmo *in itinere*, il problema regionale, che non può fare a meno di affrontare, una volta per tutte, la questione della Palestina e dei territori occupati e della strategia continuamente perseguita da Israele dell'uso della forza in quei territori, e anche il punto di vista macroregionale - ha detto molto bene il collega Tonini - con il coinvolgere nel tavolo della trattativa Siria e Iran e Iran e fare in modo che, una volta per tutte, questa area venga del tutto stabilizzata nel rispetto dei diritti dei popoli e della legalità internazionale, lasciando forse da parte le dominazioni come il grande Medio Oriente che appartengono ad altre correnti di pensiero. L'altra questione che ci preme riguarda il rilancio dell'iniziativa civile; la diplomazia per noi ha un senso se è multiforme: diplomazia degli Stati, dei Governi e diplomazia dal basso, quella cooperazione tra popolo e popolo, che il nostro Paese ha saputo conoscere, anche in maniera innovativa, durante la crisi dei Balcani, che continua a essere attiva e feconda in Iraq, in Afghanistan ed è poco conosciuta ai più, ma che ha pari dignità, secondo il nostro parere, per la costruzione di una politica estera di pace e di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti. conflitti. Accanto all'ipotesi, che noi auspichiamo una volta che la Conferenza internazionale di pace sul Medio Oriente abbia seguito ed esito, di inviare i caschi blu anche a Gaza e in Cisgiordania, ci auguriamo che il Governo italiano si impegni per la costruzione di corpi civili di pace, di strutture civili che possano andare nei territori colpiti dalle guerre, lavorare a stretto contatto con le comunità locali e ricostruire le condizioni e le precondizioni necessarie per una convivenza pacifica e, nel caso Libano, con tutta probabilità, anche prosciugando quel brodo di coltura nel quale Hezbollah rischia comunque di continuare ad avere una forte forza e preponderanza e possa essere rincoraggiato ad usare anche lo strumento militare. nostro è un ordine del giorno che recepisce anche le istanze che provengono da ampie fette del movimento pacifista, che oggi magari non scende in piazza perché sta già lavorando alla pace costruttivamente e attivamente, incontrandosi in Libano con i movimenti sociali e le forze sociali sane di quel Paese. sta cercando di comprendere come intervenire in maniera costruttiva, sostenendo uno sforzo di pacificazione che non deve essere, a mio parere, soltanto un elemento di trionfalismo di un Governo o di un altro, ma deve essere fatto soprattutto nel rispetto dei diritti di quei popoli che troppo hanno sofferto.

Signor Presidente, colleghi, prendo atto con soddisfazione che, dopo una corale approvazione, a caldo, di questa manovra, da parte di quasi tutta l'Aula, oggi iniziamo a percepire qualche

non è assolutamente cambiata: viceversa, eravamo critici allora e lo siamo forse ancora di più oggi. Il 18 agosto, infatti, siamo stati chiamati ad approvare, con urgenza, una risoluzione che allora definimmo pasticciata. Si distingueva in punti: ebbene, noi potevamo anche condividerne uno, essendo favorevoli, cioè, ad alcune iniziative per assicurare, per esempio, il sostegno umanitario alle popolazioni civili.

militare italiano presso la missione UNIFIL. Noi sosteniamo - oggi come allora - la totale indeterminatezza della risoluzione e dell'impegno italiano. Non si capiva,

la regia delle operazioni (la famosa *leadership*)? E quale l'impegno finanziario del nostro Paese in tale missione?

Nella missione libanese, invece, sono presenti soltanto sei Paesi della comunità, più altri tre (Germania, Grecia e Gran Bretagna) che hanno offerto soltanto un supporto navale.

Anche l'applicazione del codice militare di pace non sembra una misura efficiente, inviando militari su scenari di guerra: non sembra sicuramente la migliore disciplina applicabile al caso. al caso. Facendo un po' di memoria storica e riavvolgendo il nastro, ricordiamo di aver visto e sentito tutto quanto è stato detto e quanto è accaduto nelle precedenti missioni di pace,

L'ordine del giorno G4 pone il problema del rischio di riarmo delle formazioni irregolari. Dal momento che il Governo libanese ha chiesto a noi e ai Paesi che partecipano alla missione

Non possiamo non riconoscere che oggi il Governo centrale libanese non ha il pieno controllo del territorio; anzi, dobbiamo essere preoccupati perché tale Governo tollera addirittura la presenza di fazioni armate di Hezbollah che identificano Israele come la peggior minaccia per la sicurezza di quel Paese, anziché identificarla nella Siria che semmai è il Paese con quel ruolo. Dobbiamo anche pensare che il riarmo

comporti ripercussioni da parte di Israele che a questo punto si vedrebbe minacciata non soltanto da chi è in grado di controllare autonomamente ma addirittura dalle forze di intervento.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, credo che l'occasione per aprire un dibattito sul Libano, ma soprattutto per discutere di politica estera, sia un momento di grande rilievo, di grande opportunità politica. Proprio sulla politica estera, infatti, si misura la capacità di un Governo e di una maggioranza di dare sostanza alle proprie ragioni e alle proprie politiche. Signor Presidente, prima di parlare degli aspetti che riguardano la questione libanese dobbiamo soffermarci, con grande attenzione, sullo spirito che anima il Governo, la Farnesina, la diplomazia italiana, nell'affrontare questi grandi temi, che riguardano, come ci ricordava sempre il presidente Selva nella precedente legislatura, nella Presidenza della Commissione affari esteri della Camera, il futuro delle nuove generazioni. nuove generazioni. Dalla relazione e dalle audizioni nelle Commissioni Senato e Camera che più volte abbiamo svolto, mi sarei aspettato, non solo dal Ministro degli esteri ma complessivamente dagli esponenti politici del centro-sinistra, che fossero chiarite con più esattezza le posizioni sulla strategia della politica estera del nostro Paese. È chiaro, infatti, che sulle priorità noi giochiamo una grande partita. Non soltanto sulla continuità della politica estera il Parlamento è chiamato (come abbiamo fatto, più volte, noi dell'UDC) a dare dei richiami forti alla responsabilità degli uomini, delle donne, ma soprattutto dei Gruppi parlamentari, Gruppi parlamentari, ad un dovere fondamentale, quello di rispettare le regole internazionali, gli accordi presi dai nostri padri, dai Parlamenti precedenti e dai Governi che si sono succeduti, perché la continuità della politica estera non è un bene di una maggioranza: è un bene di una maggioranza: è l'intelligenza di un Paese, la memoria storica, il grande patrimonio umano che portiamo in dote non solo in Europa, ma a livello internazionale. Noi dell'UDC in più occasioni, in più contesti, lo abbiamo fatto, discutendo anche nella coalizione del centro-destra del fatto che a questo riguardo non ci poteva essere un vincolo di opportunità di maggioranza o di opposizione che legasse magari al dispetto alla maggioranza una posizione diversa da quanto sta nel codice genetico di un partito, di un atteggiamento anche storico. Noi lo abbiamo fatto, e proprio per questo abbiamo preteso coerenza politica anche da parte della maggioranza di centro-sinistra che, in alcune occasioni, vedeva in qualche modo prevalere le istanze dell'estrema sinistra, dei gruppi più oltranzisti, che prevalgono anche nello scacchiere dei ragionamenti, degli interessi che non sempre sono legati alla politica estera e quindi agli interessi del nostro Paese. Noi lo abbiamo denunciato: abbiamo detto che il Patto Atlantico era ancora un punto di riferimento importante,

che gli impegni assunti alle Nazioni Unite e nei fori internazionali dovevano rappresentare quel patrimonio culturale e politico che il nostro Paese in qualsiasi contesto nazionale e internazionale poteva portare in dote come elemento di italianità. E allora, cari colleghi senatori, il punto non è tanto confermare questa continuità per l'UDC, perché noi lo diamo per scontato, magari si tratta di riaffermarla per ricordare ad altri

Le priorità sono quelle di ristabilire una forte presenza nel Mediterraneo (e noi dell'UDC pensiamo di sì)? Pensiamo che bisognerebbe ricollegare la grande opportunità della cooperazione culturale con la cooperazione per lo sviluppo come elemento, braccio operativo, della politica estera del nostro Paese, oppure si dovrebbe lasciare tutto all'apparire, all'apparire dei nostri Ministri degli esteri, lasciando a se stessa la Farnesina, lasciando senza forniture di intelligenza e di indicazione la nostra diplomazia, lasciando ad una mera gestione particolare non solo la cooperazione culturale ma anche quella per lo sviluppo, senza ricollegarla

allora capire dal Governo e conoscere con più precisione quali sono le vostre priorità. È solo un dibattito al vostro interno, colleghi della maggioranza, per capire chi vince la battaglia tra i pacifisti più o meno veri o tra i laicisti più o meno ideologici oppure è l'azione di una parte a mio parere più evoluta di questa coalizione di centro-sinistra, che tenta di affermare la continuità della politica estera, magari nascondendo la mano? allora scoprire le carte. La nostra posizione, lo voglio dire anche agli amici del centro‑destra ma soprattutto a coloro i quali guardano alla politica con gli occhi dell'attenzione, dell'interesse nazionale, dell'interesse vero per la politica estera,

nel mondo, nello scacchiere internazionale (non dimentichiamo che l'Italia è un Paese che ha garantito con la sua presenza democrazia e pace), quando noi dell'UDC per primi abbiamo detto che su questi temi dobbiamo andare avanti abbiamo dato una mano al Paese, non certamente alla maggioranza, che non riusciva a trovare al proprio interno una coesione, lo abbiamo fatto con tale consapevolezza. Con la stessa consapevolezza ci chiediamo se c'è una maggioranza in politica estera se sui Balcani vogliamo stabilire una priorità oppure, se la priorità assoluta è quella di un grande ponte verso l'America Latina, di cui tutti parlano a parole, ma su cui nessuno investe politicamente.

avendo visitato l'America Latina qualche tempo fa, quanta attenzione c'è. Ma non è un'attenzione legata soltanto ad un sentimento verso i connazionali impegnati in quell'area, è un sentimento di interessi, cari colleghi, perché la grande tecnologia europea, unita anche alla materia prima di questi mercati, di queste straordinarie risorse, non solo dell'America Latina ma di altri continenti, può essere utile nello scacchiere delle nuove opportunità e soprattutto verso le nuove generazioni, per offrire al mercato europeo, che è sempre più esigente, non solo materia prima ma anche prodotti finiti con l'alta tecnologia europea. Se allora vogliamo parlare di questo possiamo

come se l'Italia fosse attrezzata a parlare dei massimi sistemi. Certo, siamo contenti che oggi nel Consiglio di sicurezza dell'ONU il nostro Paese può svolgere un ruolo di primaria importanza. Siamo altrettanto contenti che l'Italia possa svolgere un ruolo di mediazione anche per le questioni aperte nel Mediterraneo e soprattutto per quelle aperte in Medio Oriente, ma non è sufficiente per dire che abbiamo una politica estera. Basta un Ministro accorto come il ministro D'Alema, intelligente, oculato e che ha del suo, indipendentemente dalla casacca politica che porta, per affermare un primato di politica estera, ma non è sufficiente per il Paese la bravura di un Ministro e non è rapportabile e raccordabile alla capacità di una maggioranza di darsi una politica estera. Troppa confusione. Non dimentichiamo, Presidente, e su questo discuteremo magari in un altro contesto, ciò che sta avvenendo alla Farnesina: era il Ministero *number* *one*, il numero uno di tutti i Ministeri,

Certamente, non possiamo consentire che alcuni Sottosegretari vadano in giro per il mondo, caro vice ministro Intini, affermando che il precedente Governo ha fatto peggio della mafia in Italia. Ma dove siamo, signor Presidente? Ma vi rendete conto?

teorie, di spiegarci anche che cosa fanno le ONG, magari quelle a lui vicine, in questo Paese. Vogliamo dirci tutto o vogliamo parlare del sesso degli angeli, signor Presidente? Noi vogliamo sapere! Appoggeremo ovviamente la continuità della politica estera del nostro Paese per le ragioni a cui facevo riferimento prima, ma vogliamo sapere quali sono le vostre priorità, signor Vice Ministro: nel Mediterraneo che cosa intendete fare? Volete continuare ciò che è stato portato avanti precedentemente, aprendo un grande ponte oppure volete soltanto lasciarlo come indicazione dialettica? Nei Balcani vogliamo occuparci della ristrutturazione dopo aver mandato anche i nostri militari e mettere

del nostro ruolo in Europa, se deve essere solo quello di abbassare la testa alle scelte degli altri e relegare il nostro Paese ad un ruolo soltanto servile - gli altri producono e noi dobbiamo consumare - oppure, come ha fatto il precedente Governo, dobbiamo rinegoziare l'accordo europeo

Gasperi. Su questi temi vogliamo un confronto aperto, dialettico. Non abbiamo problemi ad affermare, noi dell'UDC prima di altri, che, sul tema della continuità, ci troverete sempre disponibili. Però questo non può essere il salvacondotto di una politica che non esiste. Nelle Commissioni, nelle sedi istituzionali, dobbiamo ritrovare la forza, il coraggio di dibattere. Dobbiamo chiarire bene, l'ho detto prima e lo ripeteremo in un documento politico nelle prossime settimane, qual è il ruolo della Farnesina e che cosa sta succedendo. Troppi cecchinaggi politici sono stati fatti, troppe scelte improprie. Abbiamo aspettato qualche mese. Adesso ce ne occuperemo, signor Presidente, e ce ne occuperemo perché non possiamo lasciare i nostri diplomatici a se stessi, perché non possiamo lasciare che alcuni membri del Governo vadano in giro per il mondo a parlare di cose inesistenti ma, soprattutto, vogliamo capire quali sono le scelte politiche che questa maggioranza vuol compiere, soprattutto usando gli straordinari mezzi di una diplomazia preventiva che anche il precedente Governo ha portato avanti.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, esprimerò un voto favorevole sulla missione italiana in Libano. Il senatore Divina dice che questo denota la nostra scarsa intelligenza, l'abbiamo sentito poco fa. Non so se sia credibile che la misurazione del nostro tasso di intelligenza arrivi dal rappresentante di un partito che ha fatto della xenofobia il proprio messaggio politico principale. In ogni caso esprimerò il voto favorevole; lo farò partendo dalla consapevolezza che quello di cui stiamo discutendo è un fatto nuovo, impossibile da confondere con le altre missioni militari, in particolare quelle in Iraq e in Afghanistan, che abbiamo fortemente contrastato nelle piazze, come movimento per la pace e in Parlamento. Chi, al contrario, mette quegli interventi sullo stesso piano opera una forzatura inaccettabile. Basta dire che la missione in Libano è sostenuta da tutte le parti in causa, Hezbollah compresi, mentre quelle in Iraq ed in Afghanistan sono fortemente contrastate dalle popolazioni locali. Oltre a ciò, non posso ugualmente condividere i toni trionfalistici usati dinanzi alla partenza delle truppe italiane per il Libano. La realtà è difficile e complessa e sarebbe un grave errore non valutarla come tale. La risoluzione 1701 è certamente un elemento positivo. Essa ha contribuito alla cessazione delle ostilità ed ha determinato anche il ritiro delle truppe israeliane dal Sud del Libano senza cedere alla richiesta israeliana del disarmo degli Hezbollah. risoluzione è giunta purtroppo in colpevole ritardo quando ormai l'invasione israeliana aveva dispiegato in pieno la propria forza distruttiva provocando terribili danni alle infrastrutture e l'uccisione di centinaia di civili. In questi giorni leggiamo sui giornali la notizia dell'esistenza di migliaia di bombe a grappolo inesplose nel Sud del Libano lasciate dall'esercito israeliano, che continuano a provocare morti e feriti, tra i quali molti bambini. La risoluzione 1701 manca di una netta distinzione tra aggressore ed aggredito. Non contiene cioè una condanna dell'intervento militare d'Israele. d'Israele. Non fa menzione della questione palestinese, vero punto di svolta di ogni politica di pace in Medio Oriente. Non c'è traccia di una semplice quanto necessaria considerazione: la pace in quella Regione sarà possibile solo quando il popolo palestinese avrà un proprio Stato. Quindi, ogni enfasi sulla capacità della missione di garantire realmente la pace è fuori luogo. Nessuno oggi è in grado di prevedere cosa accadrà nei prossimi mesi sul campo. A tutti è chiaro che la fine dell'ostilità non equivale necessariamente alla pace. Che nessuna svolta si intravede nella politica di pervicace negazione d'Israele nei confronti dei diritti del popolo palestinese. Che lo scenario politico libanese è molto fluido e complesso. La funzione politica della missione quindi assumerà contorni più definiti nel corso del suo svolgimento. E' un campo aperto ed ha diverse possibilità. Su questo deve incentrarsi il nostro lavoro: far sì che la missione svolga un effettivo compito di interposizione e di mantenimento della pace; che dia un contributo a riaprire la questione della nascita dello Stato palestinese. Quindi, la vicenda palestinese è il cuore del problema e proprio per la soluzione di questo il nostro impegno deve essere maggiormente incentrato. Ciò a partire dalla richiesta di abbattimento del muro che Israele sta costruendo per dividere i territori occupati dai palestinesi in veri e propri ghetti; dalla disdetta dello scellerato accordo militare siglato dal Governo Berlusconi con Israele che viola la nostra Costituzione, la quale esclude con nettezza accordi di carattere militare con Paesi impegnati in conflitti bellici. Non dimentichiamo che Israele ha violato ben 72 risoluzioni delle Nazioni unite. Nonostante ciò, ancora si nutre un ingiustificabile timore a schierarsi con nettezza dalla parte della causa palestinese. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, quest'estate molte voci hanno giustamente affermato che il nuovo impegno in Libano delle truppe italiane apre un importante spazio per ridiscutere la presenza in Afghanistan. Il senatore Salvi ha rilevato che la credibilità del nostro Paese in Medio Oriente aumenterebbe considerevolmente dinanzi al ritiro dallo scenario di guerra in Afghanistan. Sono molto d'accordo con queste considerazioni. Voglio dire, per essere del tutto chiaro, che se vogliamo rafforzare le considerazioni sin qui svolte dobbiamo sempre far valere il nesso tra quanto andiamo a fare in Libano e quanto ancora stiamo facendo, e dobbiamo cessare di fare, in Afghanistan. Dobbiamo far sì che un nuovo segno di pace ispiri la politica estera del nostro Governo nel suo complesso. Dobbiamo far sì che siano incontrovertibili ed evidenti a tutti le finalità radicalmente non offensive delle missioni internazionali cui il Governo Prodi ritiene di aderire e cui la maggioranza di centro-sinistra da il proprio assenso. In questo quadro l'esigenza del ritiro delle nostre truppe dall'Afghanistan è ancora più urgente di quanto non fosse prima dell'attacco israeliano contro il Libano. Senza considerare che ritirarsi dall'Afghanistan renderebbe ancora più credibile la nostra presenza in Medio Oriente nelle sue finalità di pace e gioverebbe alla sicurezza delle nostre truppe. Non mi soffermo sulla descrizione della situazione in Afghanistan che è nota a tutti. Purtroppo, anche alcuni nostri militari sono morti e altri sono rimasti feriti. In queste ore il reporter Gabriele Torsello, che speriamo venga immediatamente liberato, è tenuto in ostaggio. La produzione dell'oppio è sempre più la base del potere incontrastato dei signori della guerra. Insomma, è un disastro, al punto che lo stesso ministro D'Alema ha parlato di fallimento della missione ISAF. Dobbiamo anche riconoscere che le promesse fatte solennemente qui in Parlamento in occasione del voto sul rifinanziamento della missione lo scorso luglio sono rimaste lettera morta. Non vi è, infatti, traccia del comitato di monitoraggio che doveva servire per farci un quadro della situazione sul campo; inoltre, anche la promessa di riduzione delle nostre truppe si è dimostrata non vera.

riconosciuta come missione di pace del nostro Governo da parte delle popolazioni del Medio Oriente, deve spingerci per chiudere il capitolo della partecipazione italiana alla guerra in Afghanistan.